Onorevoli colleghi, prima di iniziare questa seduta, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in segno di lutto per le vittime dell'alluvione di Messina e di solidarietà ai feriti e alla popolazione colpita dal disastro.

Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, la commemorazione ufficiale del Senato avrà luogo subito dopo l'intervento del ministro Tremonti. il senatore Salvatore Cintola, con lettera del 29 settembre 2009, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di senatore optando per il mandato presso l'Assemblea regionale siciliana. Trattandosi di un caso di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, il Senato non può che prenderne atto. Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, autorizzo la Giunta stessa a convocarsi sin d'ora.

con la Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, presentata lo scorso 22 settembre, il Governo ha provveduto ad aggiornare le stime di crescita e il quadro di finanza pubblica per l'orizzonte temporale di previsione 2009-2013. La presentazione del documento in Consiglio dei ministri è stata

La Relazione previsionale e programmatica per il 2010, presentata contestualmente, recepisce le nuove stime e conferma la strategia di prudenza fiscale che ha guidato il Governo nel definire la politica di bilancio per il prossimo triennio. L'elevata incertezza sulle prospettive economiche, incertezza che non trova precedenti prossimi storici, ha richiesto una forte prudenza per evitare che la definizione di una manovra che impegni negli anni a venire la finanza pubblica possa produrre effetti contrari all'interesse generale. In tale orientamento è stata valutata l'opportunità di proseguire nell'opera di gestione ordinaria e prudente dei conti pubblici, in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* che sarà definita in sede europea. L'impegno in sede europea è a coordinare nel tempo le azioni comuni dei Governi. Ad oggi, a questa altezza di tempo, non c'è alcuna decisione europea in ordine alla tempistica e ai contenuti dell'*exit strategy*. È intenzione del Governo italiano mantenere questo impegno di metodo e di merito assunto da ultimo in sede ECOFIN da tutti i Paesi europei. Nel corso dell'estate 2009 le condizioni complessive e la congiuntura internazionale sono migliorate. Sono emersi alcuni segnali di stabilizzazione e poi di graduale ripresa, in particolare in Asia. I dati su questo sono esposti nella Tavola n. 1 che allegherò agli atti. Le tensioni sui mercati finanziari internazionali si sono attenuate rispetto alla fase acuta della crisi. Le Borse hanno registrato un recupero progressivo dai minimi di marzo. In ogni caso, confermiamo una valutazione espressa nelle sedi internazionali, nelle quali si parla di *tentative recovery*, un caso in cui l'aggettivo influisce in modo molto significativo sul sostantivo *recovery*. Concordiamo su queste formule e ribadiamo quanto abbiamo detto non in inglese ma in latino: siamo ancora in *terra incognita*. In linea con il miglioramento della congiuntura esterna anche l'Italia ha manifestato nei mesi più recenti alcuni segni positivi: la fiducia delle imprese e dei consumatori ha mostrato una graduale ripresa da aprile. Dallo stesso mese la produzione industriale ha arrestato la caduta, mostrando a luglio un recupero dell'1 per cento rispetto al mese precedente. Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre si è contratto dello 0,5 per cento trimestre precedente, segnando una relativa riduzione della caduta. È un po' meglio delle attese. I consumi privati hanno evidenziato un recupero rispetto al trimestre precedente per effetto anche degli incentivi per il rinnovo del parco auto, varati dal Governo nel febbraio scorso. Rilevante è stato anche, ai fini della domanda interna e del clima complessivo del Paese, l'intervento del Governo per il finanziamento degli ammortizzatori. I dati sull'andamento economico si stanno accumulando, dal traffico sulle autostrade a quello postale: tutti dati relativamente positivi. Per quanto riguarda specificatamente la finanza pubblica, si nota che l'andamento del gettito IVA al netto della componente sulle importazioni ha mostrato per la prima volta nel corrente anno un'evoluzione positiva rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il tasso di variazione trimestrale delle imposte di fabbricazione, le accise, al netto dell'imposta sul gas metano è passato da meno 2,2 del secondo trimestre al più 1 del terzo. Rispetto

Per il 2010, il miglioramento della stima di crescita del PIL rispetto al DPEF è di 0,2 punti percentuali, passando da 0,5 a 0,7 punti percentuali. Per il triennio 2011-2013, le stime di crescita del prodotto sono rimaste invariate. Tutto ciò è evidente nelle Tavole nn. 1 e 2 che allegherò agli atti. previsionale e programmatica, il Fondo monetario internazionale ha diffuso il *World Economic Outlook* di autunno, prevedendo per il biennio 2009-2010 un miglioramento sia per la crescita mondiale sia per le principali aree rispetto alle stime precedenti di luglio. Per il 2009, solo per tre Paesi del gruppo dei sette (Stati Uniti, Regno Unito e Canada), il Fondo ha previsto un lieve ribasso nelle stime di crescita; lieve perché compreso tra 0,1 e 0,2 punti percentuali. Per la Francia e la Germania, il Fondo ha previsto al rialzo le stime di crescita sia per il 2009 che per il 2010. Per il Regno Unito, la previsione al rialzo è limitata a 0,7 punti percentuali nel 2010. Anche per la Spagna le stime migliorano relativamente. Tutto ciò è contenuto nella Tavola n. 3, che allegherò agli atti. In un contesto di elevata incertezza, analoga a quella che caratterizza le economie dei Paesi più industrializzati, il Governo è stato in grado di confermare sostanzialmente gli obiettivi finanziari indicati nel DPEF 2010-2013 e di ribadire la correzione degli andamenti tendenziali dei conti pubblici a partire dal 2011. Le lievi differenze del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche rispetto al DPEF derivano principalmente dai seguenti quattro fattori: la revisione delle prospettive di crescita per il biennio 2009-2010; l'aggiornamento dei conti pubblici del 2009 in base alle attività di monitoraggio; le modifiche alla manovra di luglio introdotte in sede di approvazione parlamentare; le variazioni alla curva dei tassi di interesse. Per il 2009, l'indebitamento netto è stato confermato al 5,3 per cento del prodotto interno lordo. Il saldo sconta una ricomposizione del conto che lascia sostanzialmente invariato il livello dell'indebitamento netto in termini nominali. Vi sono infatti state variazioni compensative. La ricomposizione riflette minori entrate per 1,6 miliardi di euro, integralmente imputabili al ridimensionamento delle imposte indirette, per circa 1,5 miliardi di euro, ed a minori contributi sociali, per 0,2 miliardi Per quanto concerne le spese, le nuove stime risultano inferiori per circa 2 miliardi di euro rispetto a quanto previsto in precedenza; tale riduzione deriva dal contenimento delle spese correnti per 3,4 miliardi di euro, correlate per circa la metà a minori oneri per interessi ed all'aumento, per circa 1,5 miliardi di euro, di quelle in conto capitale. L'effetto complessivo dei fattori di variazione indicati in precedenza comporta un lieve miglioramento degli andamenti tendenziali a partire dal 2011 rispetto all'andamento delineato nel DPEF.

per effetto del diverso profilo della spesa per interessi, collocandosi a fine periodo al 2,2 per cento del prodotto interno lordo. Corrispondentemente, l'avanzo primario si riduce di 0,2 punti percentuali di PIL negli anni 2010 e 2011 di 0,1 punti percentuali nel biennio successivo, raggiungendo il 3,4 per cento del PIL nel 2013. Il debito pubblico in rapporto al PIL, in presenza di una lieve revisione al rialzo del PIL nominale, è stimato collocarsi nel 2009 al 115,1 A partire dal 2010, il debito in rapporto al PIL è previsto diminuire gradualmente, con una riduzione lievemente più accentuata di quella indicata nel DPEF, fino a raggiungere il 112,7 per cento Nel confronto con gli altri Paesi più industrializzati, secondo le stime elaborate dalle organizzazioni internazionali, l'indebitamento netto in rapporto al PIL risulta tra i più contenuti. Per essere chiari, è la prima volta in tanti anni che la velocità di crescita del deficit e del debito italiano è inferiore alla media europea. Alcuni dati indicano che molti Paesi stanno arrivando al 10 per cento del rapporto deficit-PIL. Questo comunque è un dato che non ci porta a forzare nella logica della prudenza,

l'Italia registrerebbe l'aumento cumulato di debito pubblico più basso tra i Paesi del Gruppo dei Sette, ad esclusione del Canada. Questo, ripeto, è frutto di una politica di prudenza che crediamo fondamentale continuare. La crescita del debito in Italia è principalmente spiegata dall'aumento cumulato dell'indebitamento netto e dal mancato apporto della crescita, che in condizioni cicliche normali imprime alla variazione del debito un significativo contributo negativo. Quindi, se il rapporto si deteriora è per effetto del prodotto interno lordo e non per effetto di politiche di indebitamento oltre la soglia del 5 per cento, che crediamo sarebbe non prudente e non augurabile per questo Paese superare. Il contributo e l'aggiustamento *stock* e flussi risulta nettamente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi. Nel periodo 2011-2013, sulla base di uno scenario a politiche invariate, il debito pubblico italiano registrerebbe il secondo incremento più contenuto dopo quello della Germania, e questo per noi è un dato assolutamente positivo. Il debito pubblico italiano è previsto aumentare di 7,8 punti percentuali, Il ritorno su un sentiero di crescita dovrebbe contribuire a ridurre il nostro debito di alcuni punti percentuali. Tutto questo esercizio previsionale è esposto nella Tavola n. 6. In termini strutturali, nel 2009 il saldo di bilancio si deteriora per 0,2 punti percentuali rispetto al DPEF, e ciò per effetto prevalente delle maggiori misure *una tantum*. Il percorso di risanamento riprende a partire dal 2010, dopo il peggioramento del 2008 e la lieve riduzione nel 2009. Il deficit, corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum*, risulta in progressivo ridimensionamento negli anni a seguire negli anni a seguire con una correzione cumulata di circa 1,4 punti percentuali fino al 2012. In analogia a quanto è accaduto l'anno scorso, la manovra di bilancio per il prossimo triennio è stata in parte anticipata con l'adozione, già entro l'estate, di un provvedimento normativo organico. Contestualmente al DPEF, il Governo ha infatti varato il decreto-legge n. 78 del 2009, finalizzato a combinare una duplice esigenza: fornire un primo aggiornamento della manovra finanziaria triennale approvata l'anno scorso ed imprimere slancio all'economia mantenendo il controllo dei conti pubblici. Il decreto-legge è stato approvato sostanzialmente nella sua versione iniziale, fatte salve alcune integrazioni che non hanno modificato l'impatto sull'indebitamento. Il provvedimento di luglio reperisce risorse per circa 17 miliardi negli anni 2009-2012, includendo gli effetti di anticipo all'anno in corso specificamente per effetto di misure contenute nel decreto-legge e destinate a favorire una più rapida uscita dalla recessione. Altre misure riguardano interventi urgenti e indifferibili in materia di banche, di fondi, di sisma, per il rilancio di infrastrutture e dello sviluppo per la proroga di alcuni termini legislativi. Le risorse reperite sono state indirizzate a sostenere il reddito delle famiglie con interventi sul mercato del lavoro e con il potenziamento degli ammortizzatori sociali, nonché a favorire le imprese, soprattutto attraverso la detassazione degli investimenti in macchinari ed attrezzature. Per assicurare la necessaria liquidità al sostegno del settore produttivo, è stata prevista l'accelerazione dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese; ciò in aggiunta alle risorse già rese disponibili con il provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato per il 2009. Inoltre, sono state depositate misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Il percorso così delineato con il provvedimento di luglio trova la sua naturale continuità nella legge finanziaria per il 2010 e l'aver anticipato al mese di luglio la maggior parte delle misure di finanza pubblica si è tradotto anche quest'anno in un disegno di legge finanziaria estremamente semplice, limitato a pochi articoli, in linea con il contenuto della legge di di stabilità, che è il nuovo strumento destinato a sostituire l'attuale legge finanziaria, secondo il disegno di legge di riforma delle norme di contabilità e finanza pubblica già discusso nel Senato della Repubblica e attualmente in esame alla Camera dei deputati. La legge finanziaria è stata adottata in continuità con la logica di prudenza fiscale con la quale il Governo ha agito fin dall'inizio della crisi finanziaria, individuando misure che trovano adeguata copertura nell'ambito del provvedimento stesso, e quindi con un impatto fiscale quanto più possibile neutrale. Dal lato delle entrate, gli impieghi disposti sono relativi alla proroga di alcune agevolazioni fiscali legate al recupero edilizio. Viene prorogata la detrazione IRPEF per interventi di recupero al patrimonio edilizio - è del 36 per cento - nonché per acquisti di immobili facenti parte di fabbricati ristrutturati entro il 2012 ed alienati entro il 30 giugno 2013. Coerentemente con l'attuale normativa comunitaria, si dispone che la riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui lavori di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo entri a regime e non sia più prevista solo in via transitoria. Gli interventi di parte corrente comprendono l'adeguamento ai fini ISTAT della quota assistenziale a carico dello Stato di pensioni, assegni e indennità agli invalidi, attuato dall'INPS mediante l'utilizzo di trasferimenti statali a favore di INPS già previsti per altri interventi e non risultati utilizzati in sede di consuntivo INPS per il 2008. In quanto mere regolazioni di effetti contabili, tali interventi non incidono sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Viene inoltre prorogata la vigente normativa in tema di modalità di contribuzione di università e altri enti di ricerca alla determinazione del fabbisogno complessivo del settore pubblico. Vengono, infine, individuati gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nel triennio 2010-2012 nonché i relativi oneri contributivi ai fini IRAP del settore pubblico statale e vengono confermati quelli del settore pubblico non statale, università e ASL, da finanziare mediante eventuali risparmi gestionali derivanti da azioni di riorganizzazione e razionalizzazione del personale delle amministrazioni stesse. L'estensione al 2010 della facoltà di rimodulazione delle risorse dei Ministeri a favore di programmi prioritari all'interno di una stessa missione contribuirà a garantire una gestione più flessibile del bilancio dello Stato e il controllo dell'andamento dei saldi di finanza pubblica. Anche quest'anno credo possa essere dato atto al Governo di aver agito con tempestività, adeguando i tempi della politica a quelli dell'economia e della società e continuando a mantenere e a tenere in sicurezza i conti pubblici, nella convinzione che la stabilità finanziaria costituisca un fattore essenziale per il Paese e per la ripresa della crescita economica. Si tratta di un'impostazione che prosegue lungo la linea innovativa adottata per la prima volta lo scorso anno. Allo stesso tempo, la manovra così definita non circoscrive le sue potenzialità in uno spazio temporale definito ma rimette le possibilità di un suo eventuale potenziamento qualora l'emergere di maggiore gettito renda disponibili maggiori risorse finanziarie da destinare alle priorità sociali più urgenti.

causando un vero e proprio disastro ambientale, con smottamenti e valanghe di fango che hanno sommerso interi centri abitati. Ieri mi sono personalmente recato nei luoghi della tragedia e ho espresso, a nome del Senato della Repubblica, il commosso cordoglio per le vittime innocenti e i sentimenti di solidarietà e vicinanza alla popolazione così gravemente colpita. Il bilancio, peraltro ancora provvisorio, è gravissimo: 24 morti, numerosi dispersi, decine di feriti, oltre ad ingenti danni materiali e immateriali. Davanti a tale tragico bilancio, fondamentale è stato il pronto intervento dei molti soccorritori che, con grandissimo impegno e generosità, si sono prodigati per limitare gli effetti della sciagura e lenire le sofferenze delle popolazioni. Ed abbiamo assistito, in questa tragica occasione, a veri e propri episodi di eroismo. Alla Protezione civile, alle forze dell'ordine, agli operatori della Croce rossa e del Servizio sanitario e agli altri volontari rivolgo pertanto, a nome dell'Assemblea, un sincero ringraziamento. Ancora una volta il Paese piange le conseguenze di straordinari eventi calamitosi, aggravati però dall'incuria e dall'irresponsabilità umana. È ancora straziante il ricordo dell'immane tragedia che nel maggio del 1998 sconvolse la valle del Sarno, provocando la morte di 160 persone e distruggendo centinaia di abitazioni. Né possono essere rimossi dalla memoria collettiva gli altri molteplici disastri ambientali: dalle stragi del Vajont nel 1963 (in cui persero la vita 1800 persone) e della Val di Stava nel 1985, alle esondazioni dell'Arno nel 1966 e dell'Adda nel 1987, nella città di Genova nel 1970 e in Piemonte nel 1994. E a tante, tante altre devastazioni, il cui ricordo è impresso nei nostri cuori. Non è certo questo il momento di indulgere a polemiche. Piuttosto, è ora necessario uno sforzo comune per assicurare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie colpite e garantire loro la necessaria assistenza; è ora prioritario operare affinché siano prontamente realizzate nuove abitazioni da mettere a disposizione di coloro che non hanno più una casa, sulla scorta di quanto è stato realizzato per i territori abruzzesi flagellati dal recente evento sismico. È, però, impellente avviare una riflessione concreta ed operativa sulle strategie e le iniziative da intraprendere per affrontare alla radice il fenomeno del rischio idrogeologico che incombe su gran parte del Paese e per promuovere un'efficace messa in sicurezza dei territori più minacciati. Alle parole devono seguire fatti e comportamenti adeguati: lo dobbiamo a questi morti e a questa gente privata drammaticamente del proprio ambiente quotidiano. Do ora la parola al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dottor Bertolaso, che ringrazio per avere accolto l'invito della Presidenza a riferire sul tragico evento.

prima di addentrarmi nella descrizione di quello che è accaduto nella notte tra il 1° e il 2 ottobre, voglio ricordare che già pochi giorni prima del disastro di Messina (dal 25 al 27 settembre) un fenomeno meteorologico particolarmente avverso e persistente aveva già investito, oltre la Sardegna, anche la Sicilia e, in modo particolare, la Calabria ionica. In tale occasione, in Calabria si erano registrate precipitazioni per oltre 700 millimetri di pioggia, pari a poco meno della metà di quanto si registra in un intero anno nella stessa zona, determinando danni ingenti e notevoli disagi anche alla viabilità. Pure la Sicilia fu interessata dall'evento: nelle province di Palermo, Agrigento e Catania vi furono precipitazioni comprese tra i 100 e i 150 millimetri in quattro giorni, mentre la provincia di Messina fu più marginalmente colpita con precipitazioni tra i 30 e i 40 millimetri, ma con massime registrate proprio alla stazione di Santo Stefano di Briga di circa 60 millimetri e sulla quale tornerò fra poco. In quell'occasione, benché quegli eventi fossero stato segnalati come da procedure dai vari avvisi meteo e di criticità, avevo ritenuto necessario richiamare l'attenzione delle autorità locali sulla necessità di verificare per tempo l'efficacia dell'attivazione delle strutture operative e del sistema locale di protezione civile, tramite l'emanazione di un'apposita circolare contenente indicazioni operative che è stata trasmessa a tutte le prefetture e Regioni interessate il 23 settembre. Il sistema nazionale di protezione civile e il sistema d'intervento sul territorio erano stati, quindi, già sollecitati ad un'adeguata attenzione già prima degli eventi di cui parliamo oggi. Per tornare agli attuali eventi, dirò che questi ultimi sono stati generati da un sistema depressionario che proveniva dalle Baleari, che ha determinato lo sviluppo di sistemi temporaleschi particolarmente intensi nell'area del messinese. Già il 30 settembre 2009 il Servizio aveva emesso un bollettino di vigilanza meteorologica nazionale, che prevedeva per il giorno seguente diffuse precipitazioni anche a carattere di rovescio e di temporale di forte intensità sulla Sicilia. Preso atto, comunque, della difficoltà di stabilire con precisione luogo e tempo del manifestarsi di tali eventi, nello stesso giorno, alle ore 15, avevamo ritenuto prudente e necessario emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con cui si prevedevano dal primo pomeriggio del giorno successivo (1° ottobre) e per le ulteriori 24-36 ore precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità sulla Sicilia. Il successivo bollettino di criticità idrogeologica e idraulica, emesso il 30 settembre, richiamava la necessità ineludibile di attivazione di uno stato di attenzione e sorveglianza da parte degli enti locali. La Regione siciliana, infatti, dava seguito al ricevimento di questi bollettini dichiarando i relativi livelli di allerta ai sindaci interessati attraverso un proprio avviso di protezione di rischio idrogeologico. Il giorno successivo, il 1° ottobre, a seguito delle nuovi previsioni risultanti dai modelli meteorologici, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, come estensione e seguito di quello precedente, veniva emanato, con validità per le successive 36 ore, per precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. I relativi livelli di pioggia previsti, anche elevati, hanno poi portato all'emissione, alle ore 15, dello stesso giorno 1° ottobre, di un avviso di criticità per le regioni che ho citato, a decorrere dalle ore della notte e per le successive 24 ore, in cui si prevedeva anche una moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle seguenti zone di allerta: Monti peloritani e Versante tirrenico siciliano. vorrei sottolineare che al momento dell'emissione di tutti questi bollettini o avvisi le precipitazioni erano totalmente assenti sui territori orientali della Sicilia: avevano già colpito le province di Trapani e di Palermo, ma non avevano ancora iniziato ad investire la provincia di Messina. È accaduto nel tardo pomeriggio, nella notte, del 1° ottobre, con intervalli di temporale estremamente ristretti da rappresentarsi ai limiti del possibile dispiegarsi anche in corso di evento dell'azione di protezione civile. Le precipitazioni registrate nello stesso pluviometro che ho citato prima, in località Santo Stefano di Briga, frazione del Comune di Messina, dalla stazione della rete in telemisura, hanno manifestato una persistente intensità oraria delle piogge, raggiungendo il valore massimo cumulato di tale periodo di 220 millimetri. I relativi tempi di ritorno, cioè ogni tempo durante il quale si può ripetere un fenomeno del genere,

La significativa concentrazione del fenomeno è altresì rappresentata dal fatto che mentre nella stazione ubicata nel centro di Messina il valore massimo raggiunto è stato di 70 millimetri, in un comune vicino, 10 chilometri più a sud, il valore registrato è stato di 160 La Regione siciliana, come ho detto, attivava il massimo livello di vigilanza delle situazioni in atto e delle comunicazioni tra le varie componenti territoriali del Servizio di protezione civile. Tale attività di sorveglianza e vigilanza è stata guidata anche dalla consultazione del famoso PAIR - Piano per l'assetto idrogeologico regionale - che evidenziava nelle aree interessate dall'evento diverse zone classificate a rischio geomorfologico e idraulico da elevato a molto elevato, nonché dalla memoria che gli eventi, che ancora recentemente, nell'ottobre del 2007, avevano causato molti danni e disagi alla viabilità stradale e ferroviaria nelle medesime località, tra le quali Tremestieri Etneo, Alì Terme, Giampilieri, Roccalumera e Scaletta Zanclea. A seguito di quegli eventi del 25 ottobre 2007, che portarono precipitazioni intense, sempre a Santo Stefano di Briga, con circa 80 millimetri di pioggia in due ore, fu dichiarato lo stato di emergenza, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, il 21 dicembre 2007, nei Comuni della fascia ionica della Provincia di Messina. Mi preme aprire una piccola parentesi circa l'evento appena citato e le iniziative intraprese per fronteggiarlo, anche in considerazione della rilevanza che questo ha avuto nell'attuale emergenza. Gli eventi atmosferici del 2007 provocarono l'allagamento di alcuni centri abitati, frane e smottamenti, con un aumento di detriti, fango e massi, causando ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture e anche al patrimonio edilizio pubblico e privato. Con un'ordinanza, sempre del presidente del Consiglio Prodi, del 17 aprile 2008, oltre alla nomina del commissario delegato, direttore della Protezione civile della Regione siciliana, venivano disposte misure straordinarie al fine del ristoro dei danni e del ripristino delle infrastrutture di somma urgenza, nonché di studio e conseguente realizzazione di interventi strutturali di identificazione del rischio. Per tali attività vennero previsti in ordinanza, a carico della Regione siciliana che aveva dato l'intesa a questa ordinanza, 3 milioni di euro, con possibilità di utilizzare ulteriori risorse, qualora si fossero resi disponibili ulteriori 4 milioni di euro a valere sui fondi del CIPE. Ad oggi, dalle relazioni inviate al Comitato di rientro nell'ordinario, che abbiamo istituito subito dopo quell'emergenza come facciamo in questi tutti casi, risulta che il commissario delegato abbia avuto disponibilità delle prime somme solo nell'ottobre del 2008, avendo predisposto un programma di interventi per un fabbisogno complessivo che sarebbe stato comunque di 144 milioni di euro. Il commissario delegato aveva anche stabilito che tutti gli interventi indifferibili e urgenti dovessero avere inizio dal settembre del 2008. anche il sistema di attivazione dell'allertamento per quanto riguarda la situazione di possibile emergenza causata da fenomeni meteorologici e chiarire le competenze del servizio nazionale della Protezione civile e quelle affidate alle altre istituzioni. In merito all'attribuzione, onde non generare fraintendimenti, vorrei ribadire come il sistema nazionale di Protezione civile viene attivato partendo dal sistema di allertamento. È un sistema che rappresenta un insieme di procedure, che sono contenute in una direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004, adottata con la piena e totale adesione e intesa delle Regioni, che reca gli indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico a fini di protezione civile, e basate proprio su una procedura di allarmi e di segnalazioni a livello nazionale e regionale. Queste procedure vengono attuate dai centri funzionali, che sono una rete di centri operativi per il sistema di allertamento, che gestiscono tutte le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul territorio. Sulla base di un complesso sistema di valutazioni, su soglie di allerta stabilite per norma, vengono successivamente emanati gli avvisi di criticità. Al manifestarsi quindi di un evento calamitoso, l'azione di protezione civile si origina da questo sistema di allertamento e vengono attivati i piani di emergenza. Le previsioni vengono effettuate ogni mattina, tra le ore 5 e le ore 6, appena sono disponibili i modelli meteorologici, sulla base di un gruppo tecnico, cui partecipa, oltre al Dipartimento, il Servizio meteorologico dell'Aeronautica e il servizio meteorologico delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna che, in nome e per conto di tutte le Regioni, fanno le previsioni su scala sinottica su tutto il territorio nazionale. Sulla base di queste previsioni vengono poi fatte le valutazioni su scala regionale, prima, e poi, restringendo sempre più il campo, su 127 zone di allerta. L'azione della Protezione civile quindi è una delle modalità per fronteggiare il rischio idrogeologico del nostro Paese, e comunque, da solo, questo servizio non può operare efficacemente, se contemporaneamente non viene affrontata una corretta gestione e governo del territorio. Tale governo è affidato al Ministero competente e alle Regioni, Province e Comuni, e si attua mediante la realizzazione di opere strutturali di difesa dalle frane e dalle alluvioni, ma soprattutto con una pianificazione urbanistica corretta che impedisca di costruire in aree a rischio. Per gli eventi in questione, fermo restando che ovviamente lascerò una dettagliatissima descrizione, minuto per minuto, di tutto quello che è fatto, evidenzio solo che il prefetto di Messina, di intesa con il sindaco, ha ha immediatamente attivato l'unità di crisi presso la propria sede nel momento in cui giungevano le prime notizie di quello che stava accadendo e per raccordare le prime operazioni di soccorso, iniziate sin dalle prime ore della sera di giovedì 1° ottobre. Le attività iniziali si sono ovviamente incentrate nell'operazione per aprire percorsi accessibili che potessero consentire l'intervento di ricerca e soccorso e, se del caso, di evacuazione della popolazione. Il Dipartimento della protezione civile nazionale, che ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione, ha prima mandato sul posto una *task force* composta da cinque nostri tecnici esperti nel settore, per supportare gli enti supportare gli enti territoriali e locali nella strutturazione di intervento coordinato nonché per valutare la situazione del rischio ancora in atto. Successivamente, nella prima mattina del 2 ottobre, io stesso mi sono recato a Messina, prima per presiedere una riunione di coordinamento dell'unità di crisi in prefettura e poi per coordinare direttamente i soccorsi nella zona interessata dal fenomeno. Il primo obiettivo è stato ovviamente quello di consentire il raggiungimento di quelle frazioni che già dai primi momenti risultavano isolate, predisponendo anche un'area all'interno di un complesso sportivo a Briga Marina per l'impiego dei mezzi per la gestione dei materiali.

È anche stato organizzato l'intervento delle Capitanerie di porto che, oltre a pattugliare, hanno anche garantito attività di soccorso e di allontanamento delle persone ferite dagli arenili, dove avevano trovato rifugio dagli eventi in atto.

Essendo sul posto, ed essendo riunito il Consiglio dei Ministri, informavo direttamente il Presidente del Consiglio di quanto stava accadendo. Pertanto, il Consiglio dei ministri, già alle ore 9 del mattino del 2 ottobre, poteva dichiarare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, proprio per le intense ed eccezionali avversità atmosferiche che si stavano ancora verificando sul territorio della Provincia di Messina. La relativa ordinanza di protezione civile, che deve normare l'organizzazione delle attività di soccorso, di ricostruzione e di ripristino delle condizioni di normalità, è già stata predisposta dall'ufficio giuridico del Dipartimento e domani pomeriggio verrà discussa in un'apposita riunione con il Governo regionale, per definire contenuti e modalità di azione. Il Presidente del Consiglio ha già annunciato domenica, durante il suo sopralluogo a Messina che, come d'abitudine, il Presidente della Regione siciliana assumerà l'incarico di Commissario straordinario per la gestione dell'evento e i sindaci interessati avranno la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli interventi nei territori di loro competenza. Da questa mattina, il Centro di coordinamento dei soccorsi, presieduto dal prefetto, è assistito da un centro operativo interforze - insediatosi sempre in prefettura - diretto dal responsabile della Protezione civile della Regione autonoma siciliana, che coordina tutte le attività che devono essere portate avanti nel corso dei prossimi giorni per quanto riguarda l'assistenza alle persone. impiegato nelle operazioni di soccorso un numero davvero considerevole di soccorritori e di personale appartenente a vario titolo alla Protezione civile. Signor Presidente, sono 2.386 le donne e gli uomini dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Capitaneria di porto, della Regione siciliana, della Provincia e del Comune di Messina, delle Polizie municipali, del 118, della Croce rossa, dell'ANAS, delle Ferrovie, dell'ENEL e della Telecom che stanno lavorando, direi senza un minuto di tregua, sul luogo dell'emergenza, impiegando oltre 560 mezzi, fra pale meccaniche, camion ed

avendo già recuperato i quattro corpi, il numero effettivo dei dispersi accertati è di 10. Conosciamo ovviamente il nome e il cognome, sappiamo dove dovrebbero trovarsi queste altre dieci persone. L'intervento dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di tutte le altre componenti è anche mirato a cercare di trovare queste persone disperse nelle varie situazioni. il numero che appare essere in questo momento il più realistico per un bilancio pressoché definitivo di questa tragedia dovrebbe essere pari a 35 persone, considerando che ho ragione di ho ragione di credere che i dieci dispersi non abbiano più nessuna speranza di essere ritrovati in vita. Si parla di alcuni extracomunitari che potrebbero essere stati coinvolti dalla tragedia, ma mancano completamente riferimenti e informazioni al riguardo. Pertanto, noi ci basiamo ovviamente sulle informazioni che abbiamo ricevuto per poter dare delle indicazioni precise e attendibili. Mi avvio a concludere, signor Presidente. Ancora una volta debbo dar conto al Parlamento di una catastrofe, delle sue dinamiche e di ciò che è stato fatto per far fronte all'emergenza. Ho citato ancora una volta date e orari, numeri relativi alle forze mobilitate dalla Protezione civile, nomi e sigle di strutture e soggetti istituzionali, nazionali e regionali. Ancora una volta sono qui oggi per dire che, a mio modesto avviso, il Servizio nazionale della protezione civile ha funzionato, dando prova di una solida capacità di mobilitazione e di intervento, ma ancora una volta sono qui a parlare di morti, feriti, senzatetto e di vittime di un disastro rimaste senza nulla e per il momento prive di futuro. Sappiamo da sempre che l'Italia vanta il record dei rischi naturali - da quello vulcanico a quello sismico e a quello del dissesto idrogeologico - ma sappiamo anche che tali rischi sono stati sovente sottovalutati e vissuti addirittura come un ostacolo considerato ingiusto allo sviluppo delle città, delle aree industriali e commerciali, delle infrastrutture e, soprattutto, all'attività di costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Si è costruito, semplicemente, si è utilizzato il territorio come se tali rischi non fossero esistenti e non costituissero una reale minaccia alla vita dei cittadini. Nessuno può dire che la mia personale denuncia contro l'abusivismo, non certo formulata oggi per la prima volta, non abbia un fondamento documentale. Non credo di essere più informato dei fatti rispetto a quanti leggono i documenti che riguardano l'uso e l'abuso del territorio che è stato fatto in Italia. Non ho fonti personali inaccessibili ai normali lettori dei quotidiani e a quanti si sono dati la pena di leggere le relazioni, i rapporti, i risultati di una serie infinita di studi e ricerche sullo stato di salute del nostro territorio, nonché le mappe delle diverse tipologie di rischio, che evidenziano come la quasi totalità del nostro Paese vive rischi che sono anche di tipo diverso e che minacciano da più fronti gli abitanti di numerosi comuni. giusto per non andare lontano - oltre che soggetta a rischio idrogeologico, è anche il simbolo del rischio sismico del nostro Paese. Abbiamo visto che in questi giorni molti italiani - qualcuno anche con incarichi istituzionali - manifestano insofferenza e contrarietà nei confronti di chi ricorda che la buona manutenzione del nostro Paese non è stata una priorità, non per questo o per quel Governo, non per questa o per quella maggioranza: essa non è stata una priorità per tutti. Abbiamo costruito, siamo cresciuti e abbiamo agito secondo le logiche di una cultura della crescita e dello sviluppo che non ha preso in seria considerazione le reazioni della natura alla nostra pretesa di una sua indifferenza. Ho parlato di abusivismo come di una delle cause principali della tragedia che si è consumata in questi giorni nel Messinese. Intendo con questa parola l'abuso del territorio, le costruzioni fuori da ogni regola, da ogni logica e criterio di buonsenso, la pratica di considerare possibile costruire nel greto dei fiumi, sui versanti di colline instabili, sulle occlusioni artificiali del corso dei torrenti o in aree dove il rischio di frane è censito ed è conosciuto. L'abuso dal punto di vista giuridico può essere sanato, ma non c'è sanatoria che convinca la terra o l'acqua a modificare la normalità dei loro comportamenti. Possiamo dare agli incendi boschivi e al disboscamento il peso che vogliamo, considerare *ex ante* o *ex post* questi fenomeni come inevitabili e forse anche utili al progresso economico, ma non avremo mai a disposizione strumenti normativi e giuridici che impediscano ad una collina disboscata di diventare più fragile e più pericolosa. Dalla mattina del 6 aprile io vivo all'Aquila, salvo qualche viaggio a Roma e altre trasferte in giro per l'Italia legate a momenti di emergenza, difficili e dolorosi come a Viareggio e come a Messina nelle ultime ore. Due sono le lezioni che traggo da questa esperienza: la prima è che la denuncia dell'abuso del territorio non è più sufficiente, ma che occorre davvero prendere in seria considerazione l'esigenza di trasformare questa denuncia in un piano d'azione che riguardi tutto il Paese, da Nord a Sud e alle isole; se vogliamo reagire con civiltà alle tragedie di questi ultimi tempi, dobbiamo onorare le vittime del terremoto con un piano di messa in sicurezza delle costruzioni nelle aree a più alto rischio di eventi sismici, che ci sono ben note, e su questo, con il decreto-legge, si è cominciato a lavorare. Dobbiamo rendere giustizia, nel senso morale del termine, che riguarda tutti noi e non solo la magistratura (che fa il suo dovere con i propri tempi e le proprie procedure) alle vittime di Viareggio con un piano di intervento sulle infrastrutture critiche del Paese dobbiamo onorare le vittime di Messina con un piano serio di interventi strutturali di mitigazione del rischio da frane, alluvioni e colate di fango. Come ha detto anche il Presidente del Consiglio, dobbiamo trovare subito i soldi necessari per un grande piano di manutenzione del Paese, dobbiamo eliminare la zona grigia delle competenze fra gli enti centrali e le amministrazioni locali, in modo che cessi l'odioso gioco dello scaricabarile; dobbiamo investire in formazione, educazione e cultura del proprio territorio, che deve essere patrimonio di tutti e non terra di nessuno, dobbiamo immaginare meccanismi d'intervento più agili, sfruttare ancor di più le moderne tecnologie e definire anche un piano di assicurazioni contro le calamità che sia equo e realistico. Adesso attendiamo che la magistratura, alla quale tutti noi garantiamo la collaborazione necessaria, accerti responsabilità e colpe, è un passaggio necessario, ovviamente, in un Paese civile come l'Italia, ma non possiamo più affidare alla magistratura anche il compito di riscoprire per gli italiani che sovente è stato violato il buonsenso, che è stata cancellata la saggezza, che è stata considerata nemica la prudenza, che sono state ignorate informazioni e conoscenze che la scienza ci ha messo fra le mani. Non credo sia compito nostro ricercare i colpevoli, indagare alla ricerca di responsabilità personali, che probabilmente esistono: il nostro compito è diverso, è quello di prevedere fin dove possibile, far circolare nel più breve tempo che si può le informazioni sugli eventi che possono assumere le dimensioni della catastrofe, è nostro compito intervenire dopo un disastro per ridurre al minimo i disagi della popolazione. Abbiamo visto, anche nelle ultime ore, molte persone impegnate a dare della nostra Protezione civile una immagine che non considero rispondente al vero; l'articolazione del nostro Servizio nazionale, che prevede compiti precisi per il Dipartimento, per le Regioni e per i Comuni, è stata ridefinita al momento dell'approvazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione e risponde a criteri di solida efficacia ed è forse quello che ha avuto il coraggio di definire fino in fondo ruoli e competenze ed indicare con chiarezza la linea di comando e controllo. Non tutto si può prevedere da Roma, non tutto può essere disposto a livello nazionale. Nel caso degli eventi meteorologici abbiamo costruito un sistema di previsione e allertamento che non ha uguali in Europa; è basato però sul principio della condivisione istantanea delle informazioni e previsioni disponibili in una rete nazionale che vede presenti, coinvolti e protagonisti non solo il Dipartimento, ma soprattutto le Regioni. Nonostante questo, non disponiamo di alcun sistema che ci consenta di misurare in anticipo, con assoluta precisione, se i temporali che prevediamo saranno più intensi e disastrosi 10 chilometri più a Nord, o se le piogge supereranno le nostre aspettative 10 chilometri più a Sud di un qualsiasi riferimento geografico. Per questa ragione, la procedura in vigore contempla la trasmissione di segnalazioni alle Regioni al crescere della conoscenza di un dato fenomeno e, a cura di queste ultime, ai sindaci dei Comuni delle aree che possono essere interessate da fenomeni temporaleschi intensi. Questo nel presupposto che ciascun livello del sistema metta in campo una capacità d'azione proporzionale al rischio presente sul territorio di ciascun Comune, affidata quindi in ultima istanza all'attenzione dei sindaci e delle autorità locali, gli unici in grado di conoscere gli effetti che un temporale, anche di inusitata intensità, può avere sul proprio territorio, sapendo questi sindaci che su 24 ore al giorno, ogni minuto, ogni secondo e ogni ora, è garantita l'assistenza, la presenza e l'affiancamento del Dipartimento nazionale ai loro problemi e alle loro difficoltà. Ma se non si prende atto che le soglie di rischio presenti sul territorio si sono alzate, per l'uso e abuso che ne abbiamo fatto, e che occorre mettere mano a interventi strutturali ormai indispensabili per riportare le soglie di rischio a livelli accettabili, non potremo dire di aver tenuto conto della lezione che le recenti catastrofi ci hanno ancora una volta riproposto con forza. Signor Presidente, onorevoli senatori, deve essere ben chiaro a tutti che la natura non uccide; è l'uomo la causa delle morti che dobbiamo registrare come conseguenza di calamità naturali. Questo ripeto da anni e l'ho ripetuto anche nelle scorse ore, avendo il conforto anche della massima carica istituzionale del nostro Paese, e lo ripeto anche a me e a voi per sentirmi coerente non con il ruolo che ricopro, ma con il senso di un servitore dello Stato e delle istituzioni in un Paese che è e deve restare un esempio di civiltà anche nel saper riconoscere gli errori del passato e impegnarsi a mettere in atto le misure necessarie, non solo per non ripeterli in futuro, ma anche per dimostrare la voglia e la forza di cambiare mentalità e per l'amore che dobbiamo portare per la nostra terra. *(Applausi dai lei, signor Sottosegretario. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non è qui in discussione il sofisticatissimo sistema della Protezione civile, con il quale vengono previsti eventi che possono anche, in ragione della situazione idrogeologica del nostro Paese e del suo rischio sismico e vulcanico, condurre ad eventi e tragedie come quella che si è verificata in questi giorni. In discussione è altro: discutiamo del perché, essendo tale sistema così sofisticato nel prevederli, non riusciamo ad evitarli e perché ciò costi ogni volta tragedie con decine di morti. Quindi, la presenza del sottosegretario Bertolaso che ringrazio di essere venuto - in questo caso rappresenta la parzialità dell'approccio che questo Governo sta prestando alla materia, e non solo oggi. Sarà il passare del tempo e la capacità che avremo di chiudere definitivamente "l'età dell'innocenza", ossia di andare per davvero a individuare le responsabilità di ciascuno, che ci condurrà alla capacità di dire chi ha sbagliato, chi non è stato sufficientemente solerte, chi non ha ottemperato alle prescrizioni della circolare, chi al centro funzionale della Regione non ha avvertito i sindaci e quali sindaci non sono stati in grado in grado di valutare l'entità del rischio. Ma la verità è che su quel banco non dovrebbe esserci lei, signor Sottosegretario. Diamo come sempre atto alla Protezione civile dell'efficacia, della solerzia e della generosità con la quale si spende nell'emergenza; Governo dovremmo vedere seduti il ministro Matteoli (che si è allontanato) e il Ministro dell'ambiente. Dovremmo probabilmente avere la responsabilità anche del Presidente del Consiglio e - me lo lasci dire - del ministro Tremonti, se è vero (com'è vero)

Se dobbiamo aprire una riflessione, in questo tempo in cui ciascuno ovviamente cerca una scappatoia se è stato protagonista e magari individua nell'abusivismo una concausa importantissima dei danni che si sono verificati, dovremmo forse ricordare che nel 1994 e nel 2003 vi sono stati due condoni edilizi generalizzati e che stava per partire, anche nella mia Regione, un piano casa dagli effetti sul territorio, a nostro

stanno: le risposte un po' confuse che sono venute dal Governo in questi giorni proprio in quella terra, l'evocazione del Ponte sullo Stretto mentre sta crollando un fronte che riguarda i Peloritani e i Nebrodi (e anche la Calabria, come lei ha voluto ricordarci, sia pure tra le righe), le dichiarazioni che riguardano la necessità di spostare altrove gli insediamenti abitativi o i continui attacchi all'abusivismo e alle responsabilità dei sindaci forse ci dovrebbero indurre a guardare le cose come stanno. le cose come stanno. Per fare un esempio, soltanto in provincia di Messina abbiamo 100 frazioni collinari, quasi sempre corrispondenti ad insediamenti medievali, che sono a rischio di venire giù, tutti,

in queste ore un'interrogazione presentata allora da un collega dell'Assemblea regionale, Panarello. Era già scritto. Lei ha ricordato correttamente l'opera che il Governo Prodi mise in campo e il fatto che fino ad oggi quell'opera non ha avuto compimento. Non nascondiamoci dietro un dito. Quello che dobbiamo fare, quello che c'è da fare, è un'opera importantissima: la messa in sicurezza del territorio rispetto alle alluvioni e alle frane. Serve poi un piano di adeguamento antisismico, che era stato opportunamente previsto nel decreto sul terremoto e che invece il Governo pare si sia rimangiato. infine riportare gli stanziamenti per la difesa del suolo ai livelli che erano stati stabiliti con la finanziaria 2008. Ma, soprattutto, dobbiamo dirci la verità:

i boschi di quella zona, conta l'abbandono delle campagne, ma conta il fatto che di fronte a tutto questo non possiamo pensare di mettere dei rattoppi. Penso che non sia affatto il momento - ha ragione il Presidente della Repubblica - di evocare opere eccezionali. Ciò che dobbiamo fare è mettere con sistematicità e con caparbietà in ordine e in sicurezza il nostro territorio. Non c'è niente di straordinario da fare se non l'opera straordinaria, che è questa. Altrimenti parleremo ancora una volta di tragedie annunciate, di avvisi inascoltati, di paure dimenticate, di voci seppellite. Io invece vorrei che una volta tanto in questo Paese avessimo memoria di quello che accade! accade! L'alluvione del 2007 causò i danni che causò. Come è stato possibile consumare questa memoria nello spazio di un anno, bruciarla? Com'è stato possibile? Non è possibile bruciare continuamente ciò che accade, avere grandi momenti di commozione, le commemorazioni, la solidarietà, gli sforzi che, certo, tutti quelli che partecipano che partecipano onorano, ed essere un Paese così arretrato e sordo e dimentico ogni volta che c'è da mettere mano a un'opera che è l'unica opera possibile

alle famiglie di coloro che a Messina hanno perso la vita, e la mia vicinanza alle famiglie dei feriti e dei dispersi. Quello che è avvenuto a Messina è gravissimo, non solamente perché era prevedibile e poteva essere, almeno in parte, evitato. C'è un problema più profondo. Quella che è accaduta è solo l'ultima delle tragedie di questo genere. Nel nostro Paese abbiamo - diciamo così - la cattiva abitudine di piangere troppe volte lacrime facili, evitando invece di intervenire in via preventiva attraverso una precisa programmazione delle opere, e di destarci all'improvviso quando ormai è troppo tardi. Sull'onda delle emozioni e di alcuni inutili dibattiti in televisione si decide di varare dei provvedimenti - talvolta senza avere le risorse necessarie - e poi molte volte, dopo poche settimane, non si dà seguito a quanto previsto. Il tutto piomba così nuovamente nell'oblio. Ma la nostra storia e la conformazione del nostro territorio non consentono distrazioni, basta pensare al costo inestimabile della vita umana. Vi è la necessità di rivedere la legislazione - in parte anche quella più recente - e di riflettere molto e a lungo sulla sicurezza del nostro territorio. Penso all'opportunità di rivedere il piano casa possibilmente integrandolo in un più articolato piano di sicurezza del territorio nazionale. In Sicilia il Presidente della Regione, onorevole Raffaele Lombardo, ha già annunciato di voler rivedere il disegno di legge regionale sul piano casa, pensando bene alla possibilità di non aumentare la cubatura, specialmente in zone a rischio. Bisogna intervenire su questo, ma non solamente. Credo che si dovrebbe intervenire - anche, perché no, in funzione anticrisi - con provvedimenti che incentivino i privati ad investire in sicurezza. Si possono prevedere incentivi per chi abbandona la casa situata in luoghi a rischio idrogeologico e acquista una nuova abitazione. Credo che altre agevolazioni dovrebbero riguardare i Comuni. Dobbiamo rivedere il rapporto tra entrate e uscite degli enti locali. I Comuni che investono sulla sicurezza - prevenendo per esempio il rischio idrogeologico o altri rischi per la popolazione - dovrebbero beneficiare di deroghe al patto di stabilità. Emozione estemporanea, oblio e ancora lacrime facili: è questo - ripeto - il circolo vizioso che andrebbe una volta per tutte che Messina dovrebbe insegnarci è quello stesso che Sarno non ci ha insegnato. È ciò che - per altro verso - non ci ha insegnato nemmeno San Giuliano. Vedremo se le cose cambieranno dopo L'Aquila e Messina. Messina non è una città fortunata. Nel corso degli anni ha dovuto confrontarsi con grandi tragedie, ma anche con enormi problemi. Si pensi all'irrisolto il Governo dovrebbe pensare a mettere in campo risorse straordinarie che ridisegnino il volto di questa città, approntando un piano di edilizia che dia risposte all'emergenza, ma anche ad alcuni antichi problemi mai risolti. Sul piano operativo, sulle decisioni da prendere, vogliamo sottolineare con forza che mancano all'appello ancora diverse persone e che certamente non ci si può rassegnare a tempi lunghissimi. sappiamo infatti che il fango si sta solidificando - è necessario intervenire con ogni mezzo e con la determinazione necessaria a recuperare presto tutti i corpi. Al contempo va dato atto dello straordinario impegno dei Vigili del fuoco di tutti coloro che hanno dato soccorso in questi giorni e che ancora in queste ore si stanno adoperando per portare i soccorsi. Per quanto riguarda le fasi successive, apprezziamo le parole del Presidente del Consiglio, che ha affermato di voler prendere ad esempio il "modello L'Aquila" sia per i tempi sia per le modalità della ricostruzione. Attendiamo di conseguenza che al prossimo Consiglio dei ministri si intervenga con un apposito decreto-legge per stanziare i fondi adeguati alle necessità della ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori a rischio. Vorremo dire a tale proposito che sarebbe un buon segnale non attingere una volta tanto ai Fondi per le aree sottoutilizzate. Dobbiamo prevedere immediatamente la sospensione del pagamento delle imposte ancora dovute ed una adeguata riduzione delle stesse. In realtà non vorremmo

Non è forse anche questo un lutto nazionale? A questo proposito la scelta della FIGC - che ha autorizzato il minuto di raccoglimento soltanto per gli incontri che vedevano impegnate le squadre siciliane - è stata non solo grave, ma significativa di un clima più generale, che voglio denunciare. Credo che il problema sia complesso e riguardi direttamente anche il sistema dell'informazione, che tende a dare un diverso taglio alle tragedie che si verificano a latitudini diverse. È sembrato che i sentimenti di solidarietà e di pietà in questa occasione siano passati in secondo piano. Ci sono infatti ancora molti dispersi, però il problema sembra essere esclusivamente la caccia alle inefficienze e alle responsabilità. È sbagliato e semplicistico imputare ogni colpa ai soliti cattivi amministratori meridionali. A questo riguardo, abbiamo molto apprezzato le equilibrate affermazioni che ella, signor Sottosegretario, ha pronunciato oggi. Per altro verso ritengo - concludendo - che è stato fuorviante tirare in ballo la questione del Ponte, come se la volontà di realizzare quest'opera fosse incompatibile con la messa in sicurezza del territorio. Come se, in altre parole, in Sicilia, come in altre Regioni del Sud, ci sia imposto di scegliere tra sicurezza Penso che il Governo sarà molto sensibile e che si potranno fare entrambe le cose. Signor Presidente, nella notte tra giovedì e venerdì scorso un ciclone extratropicale ha scaricato su Messina e su Scaletta Zanclea circa 220 millimetri di pioggia in cinque ore. Per cinque ore consecutive quei territori, in particolare i villaggi della zona sud della nostra città ed il comune di Scaletta, sono stati martellati da vere e proprie bombe d'acqua. Siamo in presenza di un evento eccezionale, che si verifica una volta ogni 200 anni. Le diamo volentieri atto, signor Sottosegretario, e diamo atto all'intero sistema della Protezione civile, di avere prodotto lo sforzo massimo nel tempo più breve possibile. Siamo sinceramente riconoscenti ai Vigili del fuoco, a tutte le forze dell'ordine, all'Esercito, al personale della Provincia e del Comune di Messina, all'università e alle tantissime associazioni di volontariato per ciò che hanno fatto e stanno facendo. al Corpo forestale regionale, senza la cui esperienza sarebbe stato molto più difficile accedere ai luoghi della frana, e agli stagionali della Forestale (i "centogiornisti"), che conoscono palmo a palmo la vallata di Giampilieri e che si sono resi particolarmente utili nelle ricerche, con buona pace di quanti si ostinano a chiamarli in senso dispregiativo precari. Mi consenta di esprimere un sentimento speciale di gratitudine ai tanti cittadini messinesi che sono scesi in strada mettendosi a disposizione dei centri di raccolta, delle strutture alberghiere che ospitano gli sfollati e di chiunque avesse bisogno. la compostezza e la dignità dei familiari delle vittime e i piccoli e grandi gesti di eroismo, come quelli di Simone Neri e di tanti altri, che meritano

Non mi iscrivo, quindi, al gioco di pessimo gusto su chi ha segnalato prima e che cosa e chi ha fatto prima e che cosa. Non sarebbe giusto, soprattutto per rispetto delle vittime e dei loro familiari, alcuni dei quali a me particolarmente cari. Credo che le parole più giuste e più obiettive per descrivere questa immane tragedia le abbia usate un giornalista del «Corriere della Sera», definendo il disastro messinese: «Una alleanza perversa di fattori meteorologici e geologici esaltati dall'intervento umano». Prosegue il giornalista: «Le bombe d'acqua sono state l'elemento scatenante. La fragilità intrinseca dei monti del Messinese e l'imprevidenza dell'uomo hanno fatto il resto». Ma prima ancora dell'attività edilizia, la mano dell'uomo ha inciso brutalmente su quei territori con gli incendi dolosi, che hanno totalmente disboscato il suolo. L'abbandono delle colture tradizionali e della pratica dei terrazzamenti ha contribuito poi a rendere più violento il cedimento della montagna. A questo si aggiunge lo sviluppo urbanistico ed edilizio disordinato ed esagerato. Ma il territorio di cui stiamo parlando, i villaggi di Giampilieri, Altolia e Molino, non sono nati ieri e neanche avantieri. Essi fanno parte dei 48 villaggi della città che hanno resistito ai terremoti ai terremoti ed ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Sono stati il rifugio della città e ne hanno salvaguardato l'identità e l'esistenza. In quei luoghi lo sviluppo urbanistico, per la verità, è sempre stato contenuto e consentito prevalentemente ed eccezionalmente per l'edilizia popolare e residenziale pubblica, e cioè solo per chi non poteva permettersi di comprarsi una casa. La vera espansione edilizia della città non è stata lì, né lì sono state fatte le vere speculazioni edilizie. Esse sono avvenute in altre parti (le più centrali) della città e con ben altri effetti distorsivi del territorio cittadino, tutte a rischio sismico oltre che a rischio di dissesto idrogeologico.

quasi che chi è morto o chi è rimasto senza casa se la sia andata a cercare. Non è questo il tempo delle polemiche, ma non è neanche tempo di passerelle e di sciocchezze. Alcuni esponenti di questo Governo, ad esempio, hanno scelto il posto e il momento sbagliato per le loro improvvide passerelle terrestri ed aeree, lasciandosi andare ad inesattezze su finanziamenti concessi e non spesi, di cui nessuno ha traccia ad iniziative annunciate e mai concretamente assunte; a rivendicazioni di competenze e alla citazione di norme che si sconoscono e che si citano solo per fare bella figura in qualche salotto televisivo. La cosa più grave, però, è l'insopportabile insistenza con la quale si parla proprio in questi giorni del Ponte sullo Stretto. Ma come si fa, con una tragedia di tali dimensioni ancora in corso, a sostenere l'attualità o addirittura l'urgenza di questa opera faraonica? Sappiamo che non ci sono o non si trovano le risorse per fare una serie di interventi strutturali finalizzati all'attenuazione del dissesto idrogeologico. Lei, Sottosegretario, ha parlato di 25-26 miliardi di euro di cui c'è bisogno. L'ufficio del Genio civile di Messina e il Comune di Messina, senza alcun successo, hanno tempestivamente indicato una serie di interventi urgenti per tamponare i danni, per un importo di circa 18 milioni di euro, senza avere avuto la benché minima risposta né da Roma né da Palermo. Tali interventi sono stati perfino inseriti nella proposta di rielaborazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, che ha esteso le zone a rischio fotografando anticipatamente anche il dissesto delle colline di Giampilieri, di Altolia e di Molino, senza che il nuovo PAI sia stato ancora approvato in Regione - si dice - per mancanza di personale. Come si innesta un'opera di tali dimensioni in un territorio come quello messinese? Un'opera che implica un dispendio di risorse che sarebbero tutte da concentrare - sono d'accordo con lei - per bonificare il territorio. Noi siamo d'accordo con lei, signor Sottosegretario: meno feste e meno sagre per i sindaci, ma anche meno propaganda ed opere faraoniche per il Governo. Tutto ciò dovrebbe essere ovvio e rispondere alla logica del buon padre di famiglia, interpretata con disarmante semplicità dal presidente Napolitano. Porti in Aula una norma per il Comune di Messina, nel decreto-legge che state approvando, con cui si sospende l'attività edilizia nelle zone a rischio, e noi la approveremo subito. Sospendiamola fino a quando non si predisponga un piano reale ed efficace per contrastare il dissesto idrogeologico. Signor Sottosegretario, dica al Ministro delle infrastrutture che solo lo scavo di fondazione del pilone del Ponte credo abbia una profondità di circa 70 metri ed un diametro di non so quante decine di metri, ed è baricentrico ai due laghi della riserva naturale di Ganzirri che rischiano di essere prosciugati da un intervento di posa in opera mal riuscito. Chi dovrebbe garantirlo, i signori delle ecoballe? Tutto ciò oltre agli ulteriori fenomeni di dissesto e di erosione che una tale invasione può comportare sulle dorsali collinari e montane dell'intera zona nord della nostra città. al Ministro che la viabilità di cantiere del Ponte è sovrapposta per più del 70 per cento alla viabilità ordinaria della città di Messina e che quest'ultima, come lei ha avuto modo di constatare con la sua assidua ed utile presenza in città, è sottodimensionata rispetto alla popolazione, alle sue esigenze di mobilità e alle eventuali esigenze di e alle eventuali esigenze di protezione civile. Dopo la tragedia di Messina, il Ponte non può più essere una priorità. Se il Ministro delle infrastrutture lo vuole realizzare, prima garantisca i finanziamenti per mettere in sicurezza la città di Messina dal dissesto idrogeologico e poi ne riparleremo. I paesi direttamente esposti alle frane sono ancora in pericolo, perché bisogna ancora verificare se tutta la massa terrosa è scivolata via o se ci sono porzioni del territorio in equilibrio precario. Ci potrebbero essere altri pendii che non hanno ancora generato frane, ma che si trovano in una condizione di squilibrio; occorre verificare il materiale di accumulo delle frane, in quanto potrebbe rimobilizzarsi per effetto di nuove precipitazioni sotto forma di nuove colate di fango; va verificato il materiale lungo gli alvei per gli stessi motivi; va completato lo sgombero degli abitati per consentire tutte le verifiche sulle condizioni di stabilità dei versanti. Signor Sottosegretario, come lei ha avuto modo di constatare, il fenomeno che ha interessato i tre villaggi di Messina e il Comune di Scaletta non è episodico ed eccezionale: c'è un movimento franoso più ampio. Non si può spiegare diversamente la chiusura a giorni alterni, ormai da un mese, dell'autostrada Messina-Catania per continui smottamenti e frane che interessano i comuni di tutta la zona jonica del messinese. Occorre una mobilitazione più vasta di geologi e di geotecnici, per rilevare le frane e verificare la possibilità di altri collassi. Occorre attivare in via permanente la rete nazionale di esperti della materia. Questa è la vera priorità. Onorevole Bertolaso, gradiremmo molto che parlasse solo lei e, informato da lei, solo il Presidente del Consiglio. Sarebbe meglio, certamente utile e funzionale al successo degli interventi che avete in mente di mettere in campo. Avete detto che si farà come in Abruzzo. Anche qui, voglio evitare polemiche, ma fate attenzione a ciò che si promette e a ciò che non si può oggettivamente mantenere. Non voglio ricordare i servizi giornalistici apparsi oggi e quelli del «Corriere della Sera-Magazine», ma non credo sia possibile trasferire 2.000 persone dall'altra parte della città. Temo sia impossibile, oltre che inutile, anche perché ci sono altre 43 zone della città potenzialmente nelle stesse condizioni. Cosa dovremmo fare? Spostarli se - Dio non voglia - l'alluvione si verificasse di nuovo? Da ultimo, signor Sottosegretario, non commettiamo l'errore di delegare ad altri misure, interventi e decisioni che deve prendere solo lei. La regia deve essere nazionale, anche per evitare che continuino a verificarsi spettacoli indecorosi, come quello che ha riguardato i mancati interventi a Giampilieri dopo l'alluvione del 2007. A tal riguardo - e me ne vergogno - vorrei leggere (ma non lo farò) le ultime righe di una delle tante lettere del Genio civile di Messina riguardo alla situazione di Giampilieri e alla sovrapposizione di competenze con la Protezione civile.

Anche dall'opposizione intendiamo dare il nostro contributo positivo. Lavoriamo pertanto insieme con sobrietà, con serietà e con responsabilità. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato con grande attenzione ed interesse le parole del rappresentante del Governo. Il primo nostro pensiero lo vogliamo tuttavia tuttavia rivolgere ai familiari delle vittime e alla popolazione messinese investita da questa enorme tragedia, che si poteva e si doveva evitare. Ci siamo recati a Messina nei giorni scorsi per esprimere tutti loro il nostro sentimento di profondo cordoglio e di solidarietà per i lutti subiti e per le immani difficoltà che sono costretti a sopportare, ed oggi in questa Aula intendiamo solennemente rinnovare tale sentimento. Eppure, signor Presidente, lo ripetiamo: questa tragedia si poteva e si doveva evitare. Tutti sapevamo infatti dell'avvertimento rappresentato dall'alluvione del 2007, che aveva colpito la zona interessata dall'odierna catastrofe. Tutti sapevamo degli abusi edilizi e delle violenze operate dall'uomo su un territorio ad alto rischio idrogeologico. Il Presidente del Consiglio ha addirittura affermato che questo disastro era stato previsto. Non possiamo fare a meno di dire che le parole del massimo rappresentante del Governo suonano tra l'inquietante ed il beffardo. Inquietanti perché autodenunciano l'incapacità del Governo di porre in essere azioni preventive a tutela della popolazione esposta al rischio di catastrofi naturali, anche quando tali eventi sono sono non semplicemente prevedibili, ma già previsti con estrema certezza. Suonano beffarde perché costituiscono un inutile esercizio di vanagloria sulla pelle di una popolazione che ha subito perdite enormi, innanzitutto in termini di vite umane. Sentiamo pertanto il dovere di lamentare l'inadeguatezza di un Governo che, nonostante gli altisonanti annunci, si limita ad ostentare, senza nemmeno garantirla, una «sicurezza del giorno dopo» e che, vogliamo ricordarlo, si distingue per essere un campione delle sanatorie edilizie e dei condoni. Un Governo che ha cancellato da ogni documento di finanza pubblica e di programmazione economica qualsiasi intervento specificamente dedicato alla difesa del suolo dal rischio sismico e idrogeologico, settore ormai abbandonato alla incertezza e alla inadeguatezza dei finanziamenti, con una conseguente scarsissima possibilità di programmazione e verifica degli interventi. Vogliamo qui, ancora una volta, ribadire che la crescente vulnerabilità del nostro Paese è dovuta, oltre che ad eventi naturali legati a fenomeni meteorologici e climatici, anche allo scoordinato processo di urbanizzazione del suolo e, non ultimo, ad una insufficiente azione di governo del territorio e di prevenzione dei rischi idraulici e geologici. Non si è stati in grado, né si è ritenuto importante finanziare, pianificare e programmare le attività di difesa del suolo, con l'effetto di aver colpevolmente rinunciato alla logica dell'intervento ordinario preventivo e di aver invece privilegiato la logica dell'emergenza, sempre più costosa. A questo punto occorre fare luce su quanto accaduto. È urgente ed indispensabile, anzitutto, procedere all'accertamento delle responsabilità, se è vero che i tecnici della Protezione civile, nella relazione consegnata alla procura un anno fa, indicarono le scelte territoriali determinanti negli effetti nefasti provocati dal dissesto idrogeologico. È doveroso, quindi, sapere se le case travolte dal fango costituissero abusi edilizi o se fossero state autorizzate in sanatoria, se è vero che solo ora si sente il bisogno di annunciare il pugno duro contro l'abusivismo edilizio e il ritiro del disegno di legge sul cosiddetto piano case in Sicilia. Occorre sapere se, anche in presenza di autorizzazioni formalmente regolari, i controlli e le verifiche tecniche prescritte dalle leggi in materia edilizia, urbanistica ed idrogeologica fossero stati realmente compiuti inoltre, verificare se è vero che nella sola frazione di Giampilieri sarebbero stati emessi, ma non eseguiti, ben 200 ordini di demolizione di manufatti abusivi, È doveroso, quindi, sapere quali provvedimenti sono stati adottati a seguito dell'alluvione del 2007 per mettere effettivamente in sicurezza il territorio e la sua popolazione e sapere come siano stati impiegati i fondi a disposizione, sui quali occorre far chiarezza da subito. È doveroso sapere, in conclusione, quali siano le responsabilità degli enti locali, Provincia e Comune, della Regione siciliana e del Governo nazionale in tutta questa terribile tragedia. queste ragioni, per vederci chiaro e perché si affermi il principio di responsabilità secondo cui chi sbaglia deve pagare, l'Italia dei Valori ha già presentato una interrogazione urgente al Governo. Ma subito dopo i cittadini, e con loro l'Italia dei Valori, intendono sapere se e come si intenda effettivamente affrontare l'emergenza del territorio nazionale, predisponendo da subito le adeguate misure economiche, strumentali e, se necessario, normative. Nell'immediato, occorre che il Governo chiarisca come intenda riportare alla normalità la situazione in una città che ha ancora le baracche del terremoto del 1908. Ci chiediamo a questo punto, ancora una volta e con forza, che senso abbia parlare del Ponte sullo Stretto di Messina quando mancano le infrastrutture essenziali per garantire addirittura la sicurezza della popolazione che vive e lavora nelle medesime zone in cui questa inutile e costosissima opera faraonica dovrebbe insistere. Non vorremmo che ancora una volta la priorità sia costituita dagli interessi perversi a discapito delle reali esigenze dei cittadini liberi e onesti. *(Applausi Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, più che le parole in questi momenti servirebbero i silenzi. Non posso che condividere le parole del Presidente del Senato e le sue preoccupazioni. Tutto quello che noi potremmo dire fa parte di quella retorica parlamentare troppo spesso utilizzata. Quello avvenuto nella provincia di Messina è stato un disastro annunciato e oggi noi tutti siamo qui a celebrare le sue funzioni. Non abbiamo ancora seppellito i morti e mi sembra che tutto quello che potremmo dire lo diciamo a mancanza del loro rispetto.

curare questo nostro territorio cui solo noi abbiamo potuto far male e che, a volte, abbiamo potuto distruggere. Non dobbiamo dimenticare che a metà dell'800 il padano Stoppani aveva definito l'Italia «il bel Paese»;

Penso che dobbiamo investire moltissimo nell'educazione civica. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi, in particolar modo a quelli giovani, che devono amare il proprio territorio e le proprie amministrazioni.

si rivoltano contro le regole dello Stato. luogo: «Il verminaio non è ancora stato disinfestato. Il coagulo di massoneria, mafia siciliana, 'ndrangheta calabrese, borghesia politica, magistratura deviata, è ancora lì. Ed è dentro a questa supercupola che il procuratore Guido Lo Forte sta guardando», per poter risolvere il problema grave della provincia di Messina.

Ed è uno sforzo che deve fare tutto il Parlamento, non la destra o la sinistra, lo dobbiamo fare assieme per poter migliorare il nostro il nostro territorio. Abbiamo un obbligo ben preciso: dare alle popolazioni future il nostro territorio meno rovinato possibile. Non voglio fare retorica. Non conosco la situazione al di là delle immagini televisive del disastro che si è verificato. So che siamo in buone mani un Governo che ha dato prova di riuscire a risolvere i problemi, come nel caso dell'Abruzzo. Dunque, non posso far altro

nel giugno 2008 si è votato per le elezioni amministrative a Messina ed è stato eletto il nuovo sindaco. Il 27 agosto 2008, a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2007, con nota di protocollo n. 11324, il Comune ha trasmesso, su richiesta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, la richiesta di aggiornamento del PAI relativamente alla zona della Provincia di Messina, con allegato elenco delle opere per un importo complessivo di 18 milioni di euro. risultava individuato il costone di Giampilieri Superiore, a protezione del centro abitato, per un importo complessivo pari a 3,3 milioni di euro. Con nota del 27 agosto 2008, il sindaco Buzzanca inviava all'Assessorato regionale territorio e ambiente, servizio IV difesa del suolo, una relazione nella quale si chiedeva la perimetrazione di nuove aree e l'aggravamento di altre ricadenti nel Comune di Messina da inserire nel PAI regionale. Nella relazione veniva introdotta l'area di Giampilieri Superiore, che non era prevista perché il PAI era fermo al 2006.

inviava al Dipartimento generale della protezione civile di Palermo un sollecito con il quale chiedeva per Giampilieri Superiore, a seguito dell'alluvione del 25 ottobre 2007, un intervento.

Nella considerazione che gli interventi sul costone di Giampilieri Superiore erano stati avocati in capo alla Protezione civile regionale, così come previsto dall'O.P.C.M. (lo vedremo il sindaco interveniva dove gli era rimasta la competenza, cioè nei villaggi di Cumia, Santa Margherita e Torre Faro, programmando e sollecitando nuovi interventi anche in altre parti del territorio. Dico questo anche perché Buzzanca, insieme al sottoscritto, era un dirigente dei gruppi di ricerca ecologica e quindi ha ben chiaro il concetto di territorio, che è ben diverso dal terreno sul quale per cinquant'anni amministrazione e opposizione, di tutti i colori,

perché il senatore Menardi, che è un mio carissimo amico, ha scritto oggi su «Libero» un intervento nel quale sostiene che, in considerazione del fatto che la causa di ciò che è avvenuto a Messina risiede nell'abusivismo edilizio, bisognerebbe, per esempio, commissariare i responsabili degli enti locali. Certo, poveretto, cosa ha appresso dai *media* nazionali e da quanto si dice? Non certo che c'era un'amministrazione attenta che, da quando si è insediata ha cercato di capovolgere la situazione. No, ha appreso

Cosa significa "è colpa dell'abusivismo" o "incentrare i primi interventi sull'abusivismo"? Significa intanto dimenticare cosa è successo, dimenticare che si tratta di altro, e in ogni caso se c'è abusivismo vuol dire che ci sono degli abusivi. Quindi, tutto sommato, coloro che sono morti sono morti o a causa loro, se abusivi, o a causa del loro vicino, se abusivo. di una filosofia complessiva che nel caso di specie punta a punire o la classe dirigente amministrativa, contro la quale peraltro abbiamo combattuto tutti quanti per oltre quarant'anni, oppure i cittadini responsabili di tutto questo.

che i colleghi del centrosinistra si sono comportati molto meglio rispetto agli esponenti del centrodestra. I colleghi dell'opposizione hanno svolto sull'argomento interventi con un taglio completamente diverso. Certo, lo hanno utilizzato strumentalmente, lo sappiamo, per la questione del Ponte sullo Stretto, confondendo le priorità, perché un conto è la priorità sulle infrastrutture e sullo sviluppo, altro è la priorità sulla manutenzione e sul rispetto del territorio. Sono due priorità compatibili, non incompatibili, e qualche sciacallo c'è stato anche all'interno del PdL. Però, attenzione,

dichiarando lo stato di calamità naturale e il dissesto idrogeologico: siamo in una fattispecie in cui la pericolosità era già stata individuata dal Consiglio dei ministri. Lei non può venirci a dire, rispetto ad un fatto che è stato già specificato, identificato ed esattamente stabilito che c'è di mezzo l'abusivismo. No, perché un provvedimento ha già stabilito che c'è dissesto idrogeologico e che siamo di fronte ad uno stato di calamità e di pericolo.

arriva il secondo telefax, del quale lei ha parlato, in cui viene aumentato il codice di pericolosità, ma solo a cominciare dalle ore 6 del 2 ottobre e per le successive 24 ore. Cioè, quando la catastrofe era già avvenuta, la Protezione civile di Palermo

può far sentire a tutti gli italiani che quelle di Messina sono persone perbene, così come lo sono tutte le altre; che non c'entra niente l'abusivismo e che esso è un fatto di mentalità e di cultura che risale alla pratica di una classe dirigente abituata a lasciar fare,

Aggiungo che Messina non è neppure inserita nel codice R4, nonostante sia stato più volte richiesto dalla Provincia. Lei mi capisce e si rende conto di cosa intendo dire.

Sono certo che il Paese, come ha fatto nei confronti dei terremotati d'Abruzzo, saprà stringersi attorno alle famiglie e al dolore di queste persone che hanno perso familiari e la loro casa e che sono state colpite da un'immane tragedia. Non accetto l'idea che possano differenziarsi i momenti di dolore e di commiserazione: sono tutte vittime di una vicenda ecologica imprevedibile e straordinaria, e sono certo che il Paese

Nato a Genova il 1° agosto 1927, si era laureato in giurisprudenza ed era divenuto, poi, avvocato. In seguito intraprese la carriera universitaria insegnando, tra le altre, presso le università di Bari e Roma, e sviluppando un profilo di studi e interessi di respiro internazionale nelle università di Nanterre, Parigi, Los Angeles, Buenos Aires e New York. Nel 1969 divenne Presidente della Commissione nazionale per lo Statuto dei lavoratori, che ebbe 1'incarico di redigere il testo che costituisce, ancora oggi, il fondamento giuridico dei rapporti di lavoro nel nostro ordinamento. Un testo rimasto a lungo unica radice del diritto dei sindacati e dell'autonomia collettiva nel nostro frastagliato panorama normativo. Per comprendere le ragioni assurde per cui nel maggio del 1983 fu vittima di un vile attentato delle Brigate Rosse, si deve soprattutto ricordare che Gino Giugni, come in seguito Massimo D'Antona e Marco Biagi, ha rappresentato per molti anni un modello straordinario di intellettuale e giurista, alla costante ricerca di un raccordo efficace e profondo tra le più mature elaborazioni del mondo accademico e le istituzioni. In questo senso, ricordare il professor Giugni solamente come il padre della legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori, sarebbe persino riduttivo. Vale invece tornare su una sua celebre affermazione, esemplare dell'idea di riformismo e innovazione che ne ha pervaso sempre l'azione e la dottrina: «Il riformismo sociale, dal momento che non ha l'ambizione di cambiare il mondo in dieci giorni, trae alimento essenzialmente dall'osservazione empirica». Si spiega così perché egli abbia incarnato un punto di riferimento per quel diritto sindacale in divenire di cui fu, oltre che interprete, dapprima teorico tra i pionieri e poi legislatore. Dalla metà degli anni Novanta è poi Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che segnò gli esordi di quell'Autorità indipendente e ne orientò la successiva azione di indirizzo e regolazione. In ciascuna di queste vesti, i suoi contributi si sono sempre distinti per equilibrio, capacità di innovazione, sensibilità per gli interessi sociali di un Paese in costante trasformazione economica nell'arco dei tre decenni cruciali tra il 1970 e il 2000: un'inesausta missione per trasformare e ammodernare gli istituti che regolano il rapporto di lavoro, quel lavoro su cui, secondo 1'articolo 1 della Costituzione, è fondata la nostra Repubblica. Nel giugno 1983 la prima elezione a senatore nelle liste del Partito Socialista Italiano segna l'avvio di un impegno diretto nella vita politica e parlamentare italiana. Quale membro di questa Assemblea, ricoprì il ruolo di Presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale nella IX, nella X e nell'XI legislatura. Fu anche componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 e autorevole membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Nella fase di passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, dal 1993 al novembre 1994, Gino Giugni assunse l'incarico di presidente nazionale del Partito Socialista Italiano e dall'aprile del 1993 al maggio 1994 ricoprì la carica di Ministro del lavoro e della sicurezza sociale del Governo Ciampi, nell'ultimo, decisivo scorcio dell'XI legislatura. Nel 1994 fu eletto deputato e divenne membro della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera. Con Gino Giugni scompare una delle più grandi figure di giuslavorista della storia del Paese. Il suo è stato un insegnamento reso ancor più prezioso dalla non comune capacità di formare una scuola, di contribuire poi al suo consolidamento, alla formazione di decine di autorevoli giuslavoristi, alcuni dei quali hanno ricoperto ruoli di assoluto rilievo anche tra i banchi di quest'Assemblea. Ma - voglio ribadirlo - con la sua scomparsa si rinnova anche la consapevolezza di quanto bisogno abbia oggi l'Italia di uomini capaci di incidere, in un clima di ritrovata coesione sociale, non solo sui sistemi normativi, ma proprio sulle scelte di fondo che riguardano il tessuto produttivo del nostro Paese e le sue relazioni industriali. mitiga il senso della sua perdita, nella speranza che la lezione del professor Giugni continui ad essere seguita con coerenza e intensità da noi tutti e dalle nuove generazioni. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, è stato un esempio di assoluta dedizione allo Stato democratico. Incolmabile il vuoto che egli ci lascia: padre dello Statuto dei lavoratori, tenace combattente del rispetto della persona

dovrebbe essere per noi un monito ad una maggiore assunzione di responsabilità per radicare nel Paese quei grandi valori ai quali dedicò la sua vita. Voglio ricordare a questo proposito il suo appassionato lavoro per favorire la significativa stagione degli accordi. Non c'è dubbio che egli è stato uno tra i più autorevoli giuslavoristi della nostra epoca, anche se era grande la sua umiltà, tanto da attribuire i suoi meriti ai ministri Brodolini prima e Carlo Donat-Cattin dopo. Prezioso è stato il suo contributo per l'affermazione del valore della democrazia: con lo Statuto dei lavoratori la Costituzione entrò a pieno titolo e per la prima volta nelle fabbriche del nostro Paese. Quando ricordiamo Giugni dobbiamo ricordare uno studioso della lotta dei lavoratori per l'affermazione del diritto del lavoro e per la democrazia. Con lui scompare uno dei maggiori interpreti di una stagione politica e culturale che oggi appare a noi ormai lontana, una stagione in cui il dialogo e il confronto politico erano improntati all'insegna del rispetto dell'avversario, e dove cultura, ricerca della conoscenza e studio costituivano la base del dibattito e delle scelte politiche. Giugni è stato considerato il simbolo della congiunzione e della sintesi tra istituzioni, mondo economico e parti sociali, il promotore della dialettica razionale come antidoto contro le tensioni radicali. Per questo finì nel mirino delle Brigate rosse, che lo colpirono con l'intento di fermarlo, ma non ci riuscirono. Emblematico è anche il ruolo da lui svolto in quest'Aula, da senatore della Repubblica prima, e poi come Ministro del lavoro nel Governo Ciampi. Mi corre l'obbligo di ricordare altre due pietre miliari del suo lavoro: il primo accordo tripartito e la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

colleghi, è con profonda partecipazione, a titolo personale e del Gruppo dell'Italia dei Valori, che oggi intendiamo onorare in quest'Aula la figura di Gino Giugni, insigne giurista, politico attento all'evoluzione dei tempi e maestro di tante giovani generazioni. Egli è stato fautore di un riformismo ricco di contenuti, improntato all'elaborazione di programmi concreti, così diverso dalle vuote definizioni di riformismo che sentiamo in questi giorni. Il suo pensiero si ritrova in gran parte nella legislazione che, tra gli anni Settanta e Novanta, ha regolato il mercato del lavoro in Italia. Il suo essere tra i padri dello Statuto dei lavoratori (quello Statuto che molti che oggi onorano Giugni intendono addirittura smontare o colpire) ha fatto passare in secondo piano la grande importanza che Gino Giugni ha avuto come ministro del lavoro nel Governo Ciampi tra il 1993 e il 1994. In quella sede Giugni Giugni dette un contributo fondamentale a quell'accordo Confindustria-sindacati che venne descritto con un po' di enfasi - come egli stesso ammetteva - come la nuova Costituzione delle relazioni industriali. Fu indubbiamente una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera di politico, come egli stesso ricorda ne «La memoria di un riformista». Nel 1993, sotto la regia di Ciampi, tutti fecero un passo indietro, perché si resero conto che si trattava davvero di un momento epocale, in cui non ci si poteva permettere di sbagliare. Egli diceva di essere contento di esserci stato. Della validità di quell'accordo, pur ammettendo la necessità di qualche aggiornamento, e soprattutto del metodo della concertazione, rimarrà sempre uno strenuo sostenitore. Sarà fortemente critico verso tutto quello che definirà il «dialogo sociale», un metodo che riteneva inadeguato a realizzare una politica economica condivisa ed anche per questo efficace. Quando parlava del lavoro ricordava a tutti che non lo intendeva come espressione economicista. Egli intendeva il lavoro come espressione sociale e in quanto tale doveva essere difeso. difeso. Oggi vogliamo ricordare questo: in un periodo di grandi e forti tensioni occupazioni, il ricordo e soprattutto l'insegnamento di Giugni ci potrà aiutare. riconosceva nella Costituzione repubblicana una pietra miliare definitiva per il nostro Paese. repubblicana del 1948 rimarrà in vigore, noi avremo la certezza che i suoi principi etici funzionano e, soprattutto, che hanno un rilevante grado di effettività. Nel momento in cui tali fondamenti muteranno - insieme alle corrispondenti istituzioni - ci troveremo di fronte a fenomeni ai quali sarò contento di non assistere: mi auguro per per voi» - lo dice agli studenti in una lezione - «che non accadano episodi di crisi delle istituzioni tali da mettere in dubbio questi principi etici». etici». Non voglio andare oltre, perché la misura dell'uomo, la riservatezza nei comportamenti, il modo di intendere la scienza del diritto, la politica come servizio e anche la sua presenza pregnante all'interno della compagine governativa fanno di lui un riferimento che non possiamo dimenticare.

suoi allievi o addirittura suoi eredi. Dovremo cercare di essere allievi del suo pensiero, magari testimoni della nostra esperienza, in maniera puntuale al servizio del nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere ai familiari e agli amici che oggi piangono la scomparsa di Gino Giugni i sentimenti di profondo e sincero cordoglio a nome mio e del Gruppo Lega Nord, ricordiamo oggi un uomo che è stato per tutti noi un modello di vita. Da senatore, Presidente della Commissione lavoro, professore, uomo delle istituzioni, Gino Giugni non ha mai smesso di essere fino in fondo una persona vera, onesta, vorrei dire pura. Non ha mai ceduto alla tentazione della retorica, della strumentalizzazione e della furbizia. Gli interessi dei lavoratori erano per lui il faro ed il limite invalicabile per ogni proposta e politica del lavoro. In questa prospettiva non ha mai avuto paura, anzi è stato coraggioso promotore della riforma del lavoro. Gli interessi dei lavoratori non gli sono mai parsi in conflitto con l'interesse della crescita e dello sviluppo nell'intero Paese. La sua umanità era proprio la forza di saper ascoltare, comprendere e analizzare i fenomeni al di là delle apparenze, senza finzioni. La sua testimonianza è stato il suo vero insegnamento a non seguire i falsi miti di una ideologia distante dalla vita vera delle persone. Proprio la sua mitezza, il suo ragionare concreto e mai astratto, la sua tenacia nel dire sempre, con rispetto, quello che pensava rappresentavano, per chi avversava ogni progetto di riforma, una sorta di provocazione. Anche per questo subì l'aggressione vile che molti anni dopo colpì fatalmente e tragicamente altri uomini impegnati nella comune missione modernizzatrice del Paese. Penso innanzitutto a Marco Biagi e a Massimo D'Antona. Egli non fu maestro perché insegnava diritto del lavoro, ma perché testimone di quella cultura giuridica che riconosce al lavoro la dignità che permette al lavoratore di essere libero e di garantire pari libertà e dignità alla propria famiglia. I suoi percorsi sono le tracce che ancora oggi una sana politica del rispetto deve seguire per comporre conflitti, non contro qualcuno, ma a favore dell'intera collettività. Rendiamo omaggio a questa figura importantissima che, oltre ad avere ideato un nuovo rapporto tra imprese e sindacati, ha anche aperto la strada ad altre forze sindacali, fino ad allora emarginate e relegate nel ruolo di uditori dei sindacati storici tradizionali. Questo significava non emarginare le forze nuove ed emergenti, non rifiutare il contributo di tutti per il bene di tutti. Oggi noi tutti gli diciamo grazie. Grazie per la generosità di un impegno sottratto alla logica delle convenienze. Grazie per la cultura dell'inclusione di cui si è fatto interprete e garante. Grazie per quel tratto umano che è per noi tutti pedagogia del dialogo e lezione di moralità vera. Grazie, Gino Giugni, per averci saputo insegnare a raccogliere la tua lezione di umanità. Grazie, Signor Presidente, oggi abbiamo letto e sentito commemorare Gino Giugni da molti esponenti del mondo politico e sindacale. Per esempio dal ministro Brunetta sulle colonne di «Libero», dai *leader* di CGIL-CISL-UIL durante la cerimonia funebre presso la sede del CNEL e da alcuni altri. Tutti tendono a sottolineare, dell'azione di Giugni, la parte in cui trovano conferma delle proprie posizioni.

a cominciare dalla parte politica cui appartengo, a cercare con cura, nel suo pensiero, quello che mette in discussione ciascuna delle nostre posizioni in materia di politiche del lavoro e delle relazioni industriali. Il primo contributo decisivo che Gino Giugni ha dato alla maturazione del nostro diritto del lavoro e sindacale si colloca in un periodo nel quale, caduto il regime fascista e passata la bufera della guerra, l'Italia non si era ancora chiarita le idee sul come sostituire l'ordinamento corporativo. Fu Gino Giugni, con Federico Mancini, a voltar pagina rispetto all'assetto disegnato dall'articolo 39 della Costituzione, ancora essenzialmente fondato sull'idea - legata alla cultura corporativa della categoria professionale come entità definita dalla legge, alla quale il contratto collettivo avrebbe dovuto adattarsi; era l'idea fondamentale dell'inquadramento costitutivo, dominante nel ventennio precedente. Furono ancora Giugni e Mancini i primi ad affermare invece con forza l'idea che è il contratto collettivo a venire prima della categoria; è il contratto collettivo che che deve sovranamente determinare la categoria in un sistema moderno di relazioni industriali. Forse il ministro Brunetta farebbe bene a riflettere più attentamente su questa lezione

al contratto. Gino Giugni è convinto che non abbia senso cercare il diritto sindacale nel diritto statuale scritto: non certo in un codice civile lontano ormai anni luce dalla realtà del sistema delle relazioni industriali, ma neppure nella norma costituzionale, in larga parte inattuata, comunque troppo vicina, nella concezione della contrattazione collettiva a quella corporativa. Ancor meno ha senso, secondo Giugni, sforzarsi di applicare a questa materia gli strumenti della vecchia dogmatica giuridica. Egli va pertanto alla ricerca del diritto sindacale (ma anche in larga parte del diritto del rapporto individuale di lavoro) così come esso si invera nella contrattazione collettiva, nella prassi e nei rapporti che si istituiscono nel vivo del tessuto produttivo. Da questa visione del diritto del lavoro e sindacale dovremmo tutti legislatori di centrodestra e di centrosinistra, trarre motivo di ripensamento rispetto al modo ipertrofico, intrusivo, omnipervasivo, col quale siamo soliti legiferare in questa materia, "legificando"

Precursore in questa consapevolezza che la prima fonte del diritto del lavoro e del diritto sindacale va cercata non nei codici, ma nel vivo e nel concreto delle relazioni industriali, Giugni però ha sempre avuto anche una percezione molto lucida dei limiti culturali del movimento sindacale italiano. Credo che le Confederazioni sindacali maggiori farebbero bene, proprio in questo momento di commossa riflessione sulla lezione di Gino Giugni, a meditare su quanto egli ha ripetutamente detto e scritto a questo proposito. In un'intervista pubblicata nel 1992, per esempio, egli osserva che: «Il nostro è un sindacalismo... che non ha mai dimostrato un'adeguata capacità di gestione delle proprie "conquiste" anche la rivendicazione e la susseguente (eventuale) conquista contrattuale assumono importanza non tanto per il loro contenuto intrinseco, quanto per la loro capacità di creare movimento, dunque per la loro suscettibilità di costituire strumento di lotta». Giugni prosegue in quell'intervista affermando che: «Anche le grandi riforme hanno contato per il sindacato, in primo luogo, come strumento di mobilitazione. Poi, che funzionino o non funzionino affatto, o addirittura producano risultati opposti a quelli per i quali sono state rivendicate, questo importa poco; anzi: sarà occasione per invitare i lavoratori alla mobilitazione, per rivendicare la riforma della riforma». Con altrettanta lucidità Gino Giugni coglie, all'inizio degli anni Novanta, i segni dell'incipiente dualismo del mercato del lavoro e del tessuto produttivo: «La legge sui licenziamenti individuali» - egli afferma, e qui il riferimento è alla legge n. 108 del 1990 - «è un piccolo mostro che realizza in modo modesto l'obiettivo di tutelare i lavoratori delle piccole imprese, ma tutto sommato aumenta la disparità di tutela tra questi e gli altri, rafforzando la tutela nelle imprese medio-grandi più di quanto sia stata rafforzata nelle piccole: che è un vero e proprio atto di ottusità legislativa... Una riforma assai

limitava l'obbligo secco di reintegrazione ai casi di nullità del licenziamento per illiceità dei motivi, lasciando negli altri casi la facoltà di opzione per un congruo risarcimento» a ciascuna delle parti interessate. Il fatto di essere considerato il Padre dello Statuto dei lavoratori non ha mai impedito a Gino Giugni di essere fra i primi a cogliere i segni del declino del mondo in cui lo Statuto stesso era nato e a teorizzare la necessità di un adattamento ai tempi nuovi di tutto il diritto del lavoro, compresa la materia caldissima dei licenziamenti.

Signor Presidente, senatrici e senatori,

nell'opera di Gino Giugni (tutta in costruzione, in divenire, come ben spiegava egli stesso a proposito del riformismo), quelli di oggi, che forse Gino Giugni non lo ricordano, e soprattutto quelli di domani, che dovranno a lui l'aver intrapreso un cammino lungo, lento, difficile e sempre sottoposto a giudizio, che però ha garantito finora a tanti di noi noi l'opportunità di dimostrare che attraverso il lavoro le società, gli uomini e le donne si affrancano e si migliorano. Attraverso lo sviluppo del nostro Paese, di quell'alleanza che Gino Giugni interpretava forse meglio di altri e che invocava più di altri tra capitale e capitale-lavoro, egli non ha mai dimenticato che quest'ultimo è soprattutto capitale umano, è umanità. Ecco perché con Gino Giugni non muore solo uno studioso, un politico e un grande uomo, ma semplicemente muore un uomo che non ha mai smesso di amare l'Italia; un esempio da seguire per tutti coloro che sono impegnati nel difficile mestiere della modernizzazione del Paese e dei suoi sistemi. Ed è una guida che ci mancherà moltissimo: le sue idee, il suo coraggio, il suo ottimismo, la sua sobrietà, la sua capacità di essere un vero riformista ci accompagneranno sempre.

Se il riformismo non ha premesse culturali chiare, può diventare uno strumento di scambio per baratti facili, e a volte anche ineguali. Un riformismo che non sia radicato su una conoscenza del Paese e dei suoi problemi scende al basso profilo e al piccolo cabotaggio». Infatti, riformismo, per Gino Giugni, significava cambiare i principi, i criteri, i metodi della politica economica e sociale, vivificarne la cultura. Mi auguro che la sua lezione e le sue azioni ci spronino sempre a non aver paura del futuro e a non avere paura, come non ne aveva lui, di accettare la sfida di aggiornare e di modernizzazione quello Statuto dei lavoratori che forse, se oggi avesse potuto riscrivere, avrebbe chiamato Statuto dei lavori. L'impulso alla nascita dello Statuto fu dato da Giacomo Brodolini, sindacalista socialista e Ministro del lavoro, che legò il suo nome sia alla riforma della previdenza sociale che all'abolizione delle gabbie salariali.

così recita l'articolo 1 della nostra Costituzione. L'opera di Giugni ha ispirato direttamente e indirettamente, per mezzo secolo, le principali riforme del lavoro: dallo Statuto dei lavoratori, che è tuttora alla base dei diritti di chi lavora nelle imprese, al patto sociale del 1993, da lui promosso come ministro del lavoro, che ha fornito il quadro istituzionale nelle nostre relazioni industriali, alla modernizzazione del mercato del lavoro racchiusa nel patto del lavoro del 1996. Nel 1983 Giugni venne eletto senatore nelle liste socialiste e divenne, in seguito, presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale. Il 1983 è anche l'anno dell'attentato delle Brigate rosse, che inaugurarono la loro strategia

La sua lezione culturale e politica trova, a mio avviso - senatore Ichino - nel Governo Berlusconi e, in particolare, nei ministri e negli esponenti che con lui hanno condiviso storia e battaglie la più efficace traduzione e continuità. Muore uno studioso e un politico, non moriranno mai le sue idee. I giovani di allora, che con lui si sono formati nelle aule e nell'impegno politico, hanno il compito di parlare ai giovani di oggi e di trasferire loro il suo incrollabile amore per la democrazia e per la giustizia. A nome del Popolo Signor Presidente, il Governo si unisce in primo luogo alle espressioni di cordoglio che sono state rivolte da tutti gli intervenuti nei confronti della famiglia di Gino Giugni, dei suoi storici collaboratori, vicini a lui

Penso che ciò sia testimonianza di quanto egli appartenga a una memoria condivisa nel nostro Paese. È importante rilevarlo perché non sempre le sue intuizioni, le sue proposte e le battaglie nelle quali egli ha creduto sono state, nel momento in cui si sono svolte, così condivise. Il collega Ichino poco fa ha ricordato, con molta onestà intellettuale, il metodo che caratterizzava la ricerca e la proposta di Gino Giugni e alcune sue specifiche convinzioni. Io vorrei ulteriormente sottolineare quanto il suo metodo fosse quello tipico di un riformista, come è stato poco fa ricordato dalla collega Bonfrisco, cioè un metodo pragmatico seppure orientato a solidi valori di riferimento. Quel metodo lo faceva costantemente proiettato alla ricerca di efficaci punti d'incontro tra le ragioni del lavoro e le ragioni dell'impresa.

di un parlamentare alla ricerca di preferenze. Egli, senatore di prestigio in un collegio che allora si poteva considerare sicuro per il suo partito, era solito frequentare con molta curiosità le associazioni della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio, di quelle realtà produttive alle quali poco si attagliavano le relazioni industriali alle quali egli si era così tanto dedicato. La sua curiosità verso la dimensione della piccola impresa era poi rivolta all'intensità umana dei rapporti di lavoro in quelle attività produttive l'attenzione verso di esse (la cui presenza era particolarmente intensa nel suo collegio elettorale) lo portava a considerare ulteriori evoluzioni nella regolazione dei rapporti di lavoro. Ciò lo portò, per esempio, a contestare con decisione l'ipotesi (che anche allora si fece nel periodo in cui egli fu Presidente della Commissione lavoro del Senato) di estendere alla piccola impresa il noto articolo 18. Gino Giugni è certamente il padre dello Statuto dei lavoratori, cioè di quel Testo unico prodotto su richiesta del ministro Brodolini, con il quale vennero codificati norme e contratti che si erano sedimentati nel corso degli anni '50 e '60. Come ha ricordato

sapeva mettere in discussione ciò che egli stesso aveva prodotto, nella misura in cui riteneva che le condizioni fossero cambiate e che i tempi diversi richiedessero aggiustamenti, aggiornamenti e cambiamenti anche significativi. Così come egli è certamente un attore importante per l'accordo del 1993, durante il Governo Ciampi, ma, allo stesso tempo, pochi anni dopo, nel 1997, da Ministro del lavoro, istituisce una Commissione che sottopone a critica quell'accordo pure sottoscritto quattro anni prima e ne richiede una profonda modifica nella direzione possiamo dire ragionevolmente oggi - del recente nuovo modello contrattuale prodotto dalle parti sociali e condiviso dal Governo. Egli ha sempre auspicato l'unità sindacale nella modernità. Quindi, quando si è trovato di fronte alla divisione sindacale, come nel caso del patto di San Valentino, cioè dell'accordo sottoscritto il 14 febbraio 1984, pur ovviamente dispiaciuto (come tutti, allora) della mancata unità su quella misura rivolta a frenare l'odiosa tassa dell'inflazione sui salari dei lavoratori, egli non esitò poi a schierarsi e a partecipare alle tante iniziative politiche a difesa di quel patto.

parlamentare, un metodo che ha certamente influenzato molti di noi in questa Aula. Riconosco molte persone che credo possano con me dire di essere state fortemente segnate dalla vicinanza con Gino Giugni, dalla

condiviso tanti anni di militanza in quel territorio in cui egli era eletto e, come ho detto, nel quale partecipava così intensamente a tante iniziative che in quel tempo si facevano. Penso ancora al collega Maurizio Castro, con il quale nel 1988 Gino Giugni realizza un'iniziativa che mi piace spesso trovare citata con molto apprezzamento in saggi italiani e internazionali, cioè il primo Convegno dei giuslavoristi dei Paesi dell'Europa orientale, tenutosi un anno prima della caduta del Muro. un'iniziativa che ha fortemente influenzato il modo con il quale quegli stessi giuslavoristi poi sono stati protagonisti nella transizione al modello occidentale, a un sistema di relazioni industriali plurale e di tipo appunto occidentale perché ancorato all'economia di mercato e non più all'economia pianificata cui si connetteva il sindacato unico. Ho già annunciato a nome del Governo che intendiamo ricordare Gino Giugni: una prima iniziativa sarà quella di dedicare a lui uno spazio idoneo nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro, seguendo un *iter*

di Gino Giugni, che potremmo avvicinare a quello di Federico Mancini, di Marco Biagi e di Massimo D'Antona, rimanga vivo tra i tanti che vogliono continuare a coltivare quella scienza, forse non molto remunerativa dal punto di vista del reddito, ma molto remunerativa dal punto di vista della possibilità che essa offre di accompagnare quello spaccato meraviglioso delle relazioni umane che sono le relazioni industriali. Anch'io mi unisco a coloro che hanno detto: «Grazie, Gino!». la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il calendario dei lavori fino al 12 novembre. Resta confermato il calendario della settimana corrente, salvo il prolungamento della seduta odierna e della seduta pomeridiana di domani fino alle ore 20,30. Le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria - il cui esame inizierà oggi pomeriggio - dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale; gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere. Al termine della discussione sulla Nota di aggiornamento al DPEF, il Presidente renderà le comunicazioni sul contenuto del disegno di legge finanziaria. Da quel momento, con l'assegnazione dei documenti finanziari, avrà inizio la "sessione di bilancio". Le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i loro rapporti alla 5a Commissione permanente entro le ore 16 di martedì 20 ottobre. La Commissione bilancio concluderà 1'esame in sede referente entro giovedì 29 ottobre. Il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea è fissato per le ore 13 di sabato 31 ottobre. Resta confermato che nel corso della corrente settimana sarà esaminato il decreto-legge recante proroga delle elezioni a L'Aquila e che l'Assemblea non terrà seduta la prossima settimana (12-16 ottobre) in relazione ai lavori delle Commissioni per la sessione di bilancio. Nella settimana 20­-22 ottobre saranno posti all'ordine del giorno dell'Assemblea il decreto-legge recante attuazione obblighi comunitari, mozioni sollecitate dai Gruppi e ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione, fatta salva l'unanimità dei Capigruppo per quelle recanti oneri finanziari. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 21 ottobre, alle ore 12, avrà luogo la votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo in seguito alla sua elezione a sindaco di Terni. Il calendario di tale settimana potrà essere integrato con 1'esame della relazione della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, ove presentata. L'Assemblea non terrà seduta nel periodo 26-30 ottobre in concomitanza con i lavori della 5a Commissione permanente sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. La discussione dei documenti finanziari da parte dell'Assemblea avrà inizio a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 4 novembre e potrà proseguire fino a giovedì 12 novembre. I tempi sono stati ripartiti per complessive 30 ore, delle quali 18 ore per i Gruppi. Infine, la Giunta per il Regolamento sarà convocata giovedì prossimo, alle ore 12, per l'esame di proposte di modifica del Regolamento tendenti a introdurre una norma transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Sicilia, a seguito delle dimissioni del senatore Salvatore Cintola, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Sebastiano Burgaretta Aparo. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Sebastiano Burgaretta Aparo. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

al fine di dare qualche motivo di fiducia in più ai cittadini e agli imprenditori, è interessante notare l'andamento per l'anno successivo e soprattutto il differenziale rispetto alle altre Nazioni nostre concorrenti a

trarre da questa semplice analisi dei dati e dal differenziale rispetto agli anni precedenti? In sostanza, dopo la crisi, cambia nettamente lo scenario. Rimangono

non ha una sostenibilità duratura nel tempo. La seconda considerazione da fare è che diminuisce il differenziale: mentre negli anni precedenti c'era sempre un differenziale notevole tra il tasso di crescita del PIL

incentivato dall'uso del risparmio privato e quindi della crescita, che negli ultimi anni è stata notevole, di indebitamento del settore privato. fenomeno sta per finire e finisce con questo anche una crescita superiore alla norma degli altri Stati; come dire che si cresce, si cresce meno, e probabilmente questo è il tasso di crescita sostenibile.

i piedi di piombo, perché non è detto che ciò poi si traduca automaticamente in un beneficio per le economie nazionali. Banalizzando il concetto, se avessimo detassato le tredicesime investendo parecchi miliardi e poi questi fossero andati nell'acquisto di telefonini fatti in India, non avremmo fatto il bene delle nostre imprese.

Fortunatamente dal 2010 il dato torna a essere positivo, con un più 2,5, vuoi per l'effetto della detassazione dei macchinari, vuoi per l'effetto di naturale riordino delle scorte.

sul calo del PIL - quasi un terzo del PIL è fatto in esportazione, quindi va da sé che se le esportazioni cadono in questa misura i risvolti sull'economia generale sono molto importanti, non compensati da un calo dell'importazione nell'anno torna ad essere positivo il saldo importazioni-esportazioni, e questo è sicuramente un bel segnale. Permangono dubbi, a nostro modesto avviso, sul futuro andamento di inflazione e tassi di interesse. È di oggi pomeriggio il dato che, per la prima volta, il primo Stato del G20, l'Australia, torna a far crescere i tassi di interesse dal 3 al 3,25 per cento. Ciò vuol dire che, se è vero che c'è una ripartenza reale dell'economia, c'è però anche il rischio che poi ciò si traduca in un aumento dei tassi di interesse, quindi, per quanto riguarda il nostro sistema, purtroppo soprattutto del servizio del debito: un'incognita che pesa e peserà enormemente sugli anni venturi.

per gli anni venturi. Non si può di certo pensare che una finanziaria riesca ad agire sul saldo entrate-uscite, proprio perché, mentre le uscite rimangono sostanzialmente stabili, se non si incrementano

La riflessione vera da fare nei prossimi interventi di politica economica è come risolvere questo problema, che è

chiaro che siamo in grosse difficoltà. Tenuto conto che la finanziaria che inizieremo ad esaminare la settimana ventura è nell'ordine dei 3-4 miliardi - quindi nulla a che vedere con il buco entrate-uscite di 77 miliardi dell'anno venturo neanche con una delle finanziarie più corpose degli ultimi anni (la finanziaria Prodi del 2006, che era nell'ordine dei 25-30 miliardi) ci sarebbe la possibilità di

nonché contenuti aggiornamenti del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultanti da minori spese per interessi sul debito pubblico di circa 2 miliardi e minori entrate per 1,6 miliardi per imposte indirette e contributi sociali. cifre e scostamenti che non modificano il quadro dell'andamento dell'economia e dei nostri conti pubblici, tanto che per l'anno in corso e per il 2010 l'indebitamento netto viene confermato al 5,3 e al 5 per cento del PIL, mentre gli effetti sugli andamenti tendenziali producono un lieve miglioramento solo dal 2011 (lo 0,1 per cento, lo 0,2 negli anni successivi). Addirittura il saldo netto da finanziare per il 2010 risulta ulteriormente peggiorato, passando da 61,4 miliardi (dato contenuto nel DPEF di luglio) a 63 miliardi. Tutto ciò evidentemente per effetto principalmente di una sottostima del dato contenuto nel DPEF e dell'andamento incontrollato della spesa corrente, considerando anche che dall'aggiornamento delle previsioni non dovrebbero derivare effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare. Nessuna indicazione aggiuntiva di politica economica e di bilancio viene fornita rispetto a quelle contenute nel DPEF (peraltro pressoché inesistenti, come abbiamo rilevato a suo tempo), tempo), cosicché appare confermata la linea del Governo di sostanziale rinuncia ad attuare sia una politica anticiclica, che misure di correzione dei conti pubblici. I dati aggiornati che ho richiamato continuano inoltre a presentare un certo livello di inattendibilità (inattendibilità che era già stata sottolineata a suo tempo sul DPEF anche dal nostro Servizio del bilancio) se si considera, per esempio, che il Fondo monetario internazionale e l'ECOFIN non noi, l'opposizione, ma così importanti istituzioni finanziarie internazionali - qualche giorno fa, a pochi giorni dall'emanazione della Nota di aggiornamento, hanno stimato il PIL italiano in crescita per il 2010 solo dello 0,2 a fronte di una previsione contenuta nella Nota di aggiornamento che stiamo discutendo dello 0,7 per cento, con i conseguenti probabili effetti peggiorativi ulteriori sui saldi di finanza pubblica e - dato ancora più rilevante prevedendo che la disoccupazione continuerà a crescere fino a tutto il 2010 (dato di cui non si ha riscontro nelle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento), considerando anche che, come noto, l'aumento della disoccupazione incide

presenza, così come lo eravamo a luglio, della più grave recessione dal dopoguerra ad oggi. I conti pubblici hanno subito il più serio peggioramento da 18 anni ad oggi (fino al segno meno

di fronte a questo quadro drammatico e a un livello del reddito che tornerà al dato pre-crisi solo tra qualche anno, la sola linea che il Governo ha ritenuto di dover indicare al Paese, confermata qui oggi dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stata quella della prudenza, non meglio declinata: ovvero lo stare fermi in attesa che la bufera passi. È certo che la bufera passerà: ogni crisi inizia e finisce, ma, come hanno detto autorevoli economisti e osservatori, nulla sarà come prima (penso ai conti pubblici, al sistema produttivo, al mercato del lavoro e alla distribuzione del reddito). Bisognava immaginare una strategia, non solo per attenuare gli effetti sociali e finanziari della grande crisi, ma anche per governare il dopo, per immaginare l'assetto e il ruolo del nostro Paese nel mondo dopo la crisi e nella fase della della ripresa della crescita economica mondiale. Noi avevamo indicato una linea alternativa e misure precise, finanziariamente dotate, il cui baricentro era quello di agire sui consumi interni utilizzando la leva fiscale in direzione della riduzione delle imposte su redditi medio bassi e determinando, quindi, un conseguente accrescimento del reddito disponibile da utilizzare per aumentare i consumi, con tutti gli effetti conseguenti. Ci avete detto di no nel 2008, all'inizio della fase più acuta della crisi, e nei mesi successivi, fino alla discussione del DPEF di luglio scorso. Ciò lo avete fatto, come ha ripetuto oggi il Ministro dell'economia predicando, appunto, prudenza, prudenza, prudenza, e invocando solo la ripresa dell'economia mondiale. Intanto, tutti i dati della nostra economia e del nostro bilancio pubblico andavano aggravandosi in misura ed intensità

ovviamente, la posizione inerziale del Governo, mobilitata dall'unico parametro costantemente evocato, quello di stare fermi in attesa che passi e che il peggio per l'economia, per i lavoratori e i ceti deboli si attenui con gli effetti auspicati della ripresa Oggi noi riproponiamo, con la risoluzione integrativa che abbiamo depositato e con il convincimento che occorreva ed occorre più coraggio e determinazione, le nostre priorità, individuando misure che il Paese si aspetta e che configurano nel loro insieme una vera politica anticiclica. Dalla riduzione della pressione fiscale per i redditi medio-bassi al ripristino degli strumenti automatici di incentivazione delle imprese nel Mezzogiorno; dal rafforzamento degli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese alla necessità di accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione verso il sistema delle imprese, concertando uno specifico intervento con la Cassa depositi e prestiti (non riusciamo a comprendere perché almeno questa misura dal momento che la Cassa depositi e prestiti dispone di ingenti risorse liquide provenienti dal risparmio postale); dall'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno degli enti locali all'introduzione di un sistema universalistico di ammortizzatori sociali; dall'intensificazione della lotta all'evasione fiscale alla necessità di prevedere misure più incisive di controllo della spesa corrente primaria che, come è stato rilevato, è esplosa proprio in questi mesi. Signor Presidente, oggi il Ministro dell'economia, nel presentare a quest'Aula il disegno di legge finanziaria, privo di contenuti significativi, sia dal lato di una politica anticrisi e anticiclica, che da quello del controllo della spesa e dei saldi di finanza pubblica (coerentemente peraltro con l'impostazione che ho riferito sbiadita ed inefficace del DPEF), ha tentato ancora una volta di occultare il nulla della politica economica e finanziaria, dietro presunte, migliori *performance* del nostro debito pubblico in rapporto all'andamento del debito di altri Paesi. Tali affermazioni dimostrano come ancora oggi, di fronte ai dati ufficiali che si commentano da sé (il debito, come ci è noto, si attesta quest'anno al 115 per

provi a maneggiare i dati a suo piacimento per supportare questa o quell'altra argomentazione, in tal modo occultando la dura realtà di fronte al Paese. E così il debito una volta costituisce, come è stato detto più volte, per le sue enormi proporzioni, un ostacolo invalicabile per l'adozione di politiche espansive, espansive, altre volte invece viene indicato come un parametro di virtuosità rispetto a ciò che è avvenuto in altri Paesi europei. Non è vera né l'una né l'altra cosa. Era possibile ed è ancora possibile agire con la leva del bilancio, certo con prudenza, controllando e riqualificando la spesa corrente, contrastando l'evasione fiscale (è incredibile che oggi il ministro Tremonti abbia riferito di un positivo andamento del gettito IVA, come ho ascoltato e come risulterà quando invece la Nota di aggiornamento al DPEF che stiamo esaminando registra una ulteriore, corposa minore entrata allo stesso titolo), minore entrata allo stesso titolo), al fine di aiutare la nostra economia, le nostre imprese e le famiglie italiane ad uscire dal tunnel della crisi. ancora oggi a rifiutare l'utilizzo di strumenti che gran parte dei Paesi sviluppati ha adottato e il nostro Paese continua a perdere terreno rispetto agli altri Paesi europei. Noi insistiamo con la risoluzione che abbiamo presentato e ancor più lo faremo con le proposte che presenteremo durante l'esame della legge finanziaria. Fino ad oggi ci avete risposto di no, ma noi insistiamo con il convincimento che quella da noi proposta è la linea migliore per aiutare il Paese ad essere meno iniquo, più competitivo e più solido in vista della ripresa dell'economia mondiale.

rappresentano per il Paese, secondo me, un'altra occasione mancata per formulare un giudizio equilibrato sull'evoluzione della crisi e per apportare le necessarie correzioni alla politica economica e fiscale del Governo. Il Fondo monetario internazionale nel suo rapporto sull'economia mondiale formula un giudizio sintetico: la recessione globale sta finendo. Così si legge in quel rapporto. Non ha senso, a mio avviso, a fronte di questa affermazione, dividerci tra ottimisti che già assicurano che tutto tornerà presto come prima, quasi non si rendessero conto che esattamente nel «prima» si si erano create le cause del cataclisma dell'ultimo anno e mezzo, e pessimisti che guardano alla forte precarietà dei segnali di ripresa e concludono che il peggio deve ancora venire, così impedendo di vedere ciò che ha funzionato tra i molti interventi messi in atto e peggiorando ulteriormente per questa via il sistema delle aspettative. Il fatto è che l'arresto del ritmo di caduta, cioè la discreta crescita dell'economia mondiale, comunque ad un livello di quattro punti inferiore rispetto a quello pre-crisi, è frutto di una sorta di operazione aritmetica: aritmetica: una forte accelerazione dei Paesi emergenti, come la Cina, che nel 2009 è attesa realizzare un prodotto che cresce dell'8,5 per con un prodotto che crescerà del 5,4 per cento, convive infatti con la stabilizzazione ai bassissimi livelli raggiunti nei mesi scorsi da Stati Uniti d'America, Giappone ed Europa. Ci sarebbe da chiedere a quanti, tra cui il nostro Ministro dell'economia, meno di due anni fa vedevano nell'ingresso nella globalizzazione dei Paesi emergenti il principale fattore di rischio, di riconoscere oggi finalmente l'errore, ora che fanno parte anche loro della schiera di quanti vedono in una strategia lungimirante della Cina uno dei fattori essenziali del ritorno dell'economia mondiale ad una crescita soddisfacente. è un bene che l'andamento del prodotto sia tornato positivo, che le borse abbiano ripreso a salire e che le banche, salvate dall'intervento dello Stato che ha fornito loro, a spese dei contribuenti, una sorta di garanzia di ultima istanza contro il rischio di fallimento, abbiano ricominciato a fare profitti, ma assieme a questi elementi di sicuro recupero, che non ha alcun senso sottovalutare, dobbiamo considerare la sicura caduta dell'occupazione che ancora ci aspetta. Questo elemento ci fa prevedere per i prossimi mesi un possibile, anzi probabile, accrescimento dei divari sociali interni a ciascun Paese: quelli che non dispongono di un lavoro - e quindi di un reddito - saranno certamente più numerosi nel prossimo anno di quanto non siano stati nel corso dell'anno che ci sta alle spalle. È un robusto campanello d'allarme circa la solidità della possibile ripresa. Non è solo questione, colleghi, di giustizia sociale, che pure c'è e conta molto, almeno ai nostri occhi. È una questione direttamente economica. Per comprenderlo bisogna tornare sulle cause profonde della crisi: la più importante va rintracciata nell'accrescersi progressivo, nel corso di quest'ultimo quarto di secolo, dei divari di reddito disponibile fra quell'1 per cento della popolazione così ricco da poterne spendere solo una piccola parte, e quello della vasta area del mondo del lavoro dipendente autonomo collocabile nella classe media e medio-bassa. Non è un caso che la crisi sia nata negli Stati Uniti, dove questo divario si era più accresciuto nel corso degli ultimi vent'anni. Per consentire a questa enorme massa di famiglie di consumare beni molto al di là del loro reddito, reddito, la FED (Banca centrale americana) ha adottato una politica monetaria lassista. Il sistema finanziario ha inventato prodotti che, dietro la promessa della limitazione o addirittura della eliminazione del rischio, diffondevano squilibri crescenti del sistema; gli Stati Uniti hanno importato merci e capitali da paesi, come la Cina, che avevano imparato nella crisi di metà anni '90 a garantirsi da soli con un eccesso di risparmio. Quando la bolla dei valori immobiliari, posta a precaria garanzia di questa economia fondata sul debito ha cominciato a sgonfiarsi, l'intero castello è crollato. Ma in origine fu la crescita delle diseguaglianze interne; poi è venuto tutto il resto. Se è così, e a me pare che sia così, nessuna fuoriuscita dalla crisi potrà risultare sostenibile se a scala globale ed in ogni singolo Stato non verrà affrontato il nodo di un riequilibrio sociale di una relativa riduzione delle diseguaglianze. Questa strada, perseguita da ciascun Paese secondo le sue peculiarità, potrà riportarci sul terreno dello sviluppo sostenibile. E infatti lungo questo indirizzo di fondo quasi tutti i grandi Paesi si stanno muovendo, subito con politiche di bilancio duramente espansive a compensazione del collasso dei consumi interni, e con riforme di tipo strutturale, dalla *green economy* alla riforma sanitaria, come ci insegna l'amministrazione Obama. signor Vice Ministro, nelle decisioni di finanza e di politica economica del Governo italiano non c'è traccia, con il risultato che non si capisce né quale sia la ragione per la quale, anche in questi ultimi due anni, abbiamo fatto peggio della mediocre media europea, né quali siano i fattori che conferiscono credibilità alle ipotesi, che pure avanzate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, di crescita del 2 per cento l'anno per il 2011 e per tutti gli anni successivi. Dove sono gli interventi volti a favorire l'innalzamento tra un anno del prodotto potenziale? Su cosa possiamo ragionevolmente fondare una crescita così significativa in così poco tempo e per un periodo così lungo? Il Documento di programmazione economico-finanziaria, con la Nota di aggiornamento, non ci dà alcuna risposta, anzi non contiene neppure la domanda. Certo che esistono i punti di forza dell'economia italiana cui il Governo fa riferimento (un elevato risparmio privato ed un forte settore manifatturiero orientato all'esportazione), ma se il debito pubblico torna crescere trainato dalla spesa corrente primaria, del tutto fuori controllo, signor Vice Ministro, a poco varrà dal punto di vista sistemico lo sforzo di un popolo che ieri risparmiava per fiducia nel futuro - i nostri figli vivranno meglio di noi - e oggi risparmia per insicurezza e per paura del futuro. Chi comprerà nel mondo le merci dei paesi esportatori come il nostro, visto che sulla Luna forse c'è l'acqua, come ci hanno detto gli scienziati, ma ma di sicuro non ci sono, almeno per ora, consumatori che apprezzino il *made in Italy*? Non dobbiamo infatti dimenticare che nel globo esportazioni ed importazioni si debbono bilanciare nel Paese che ha fatto da consumatore mondiale nel corso degli ultimi 15 anni è ora in corso un robusto processo di deindebitamento delle famiglie. Ciò che noi critichiamo in fin dei conti è l'assoluta mancanza di ambizioni della politica economica e di bilancio del Governo. Provo quindi a proporvi i termini di una possibile svolta, coerente con l'analisi della crisi che ho appena illustrato. Primo: per crescere stabilmente al 2 per cento dal 2011 bisogna, ora, favorire un deciso innalzamento della domanda interna. Le esportazioni non bastano: quindi più spesa in conto capitale per gli enti locali - è tragicamente banale in queste ore fissare l'obiettivo prioritario del risanamento territoriale - e meno pressione fiscale sui redditi medio-bassi. Non la detassazione della tredicesima, ma tagli del prelievo permanenti che inducono al consumo e migliorano le aspettative delle famiglie. In secondo luogo, subito, interventi per aprire i mercati chiusi. Possibile che sia necessario che si muova un fondo d'investimento americano per spiegarci che con la separazione proprietaria di SNAM Rete Gas dall'ENI ci guadagnerebbero consumatori, risparmiatori e Stato? Ma allora perché non si fa? Perché non si fa immediatamente? luogo, subito le misure di riduzione della spesa corrente primaria che, adottate oggi e realizzate nel 2012, possono garantire al nostro Paese di percorrere con piede sicuro quel sentiero strettissimo che sta tra un irrigidimento della politica monetaria da parte della BCE ed una brusca svolta per un rientro dei deficit pubblici da parte dei Governi. Due scelte entrambe capaci, alla dimensione globale, di gelare sul nascere i timidi germogli di ripresa in un Paese come l'Italia nel quale il Governo, unico nel mondo, si è ostinatamente rifiutato di usare la leva del bilancio pubblico in chiave anticiclica. Certo che siamo, nel 2009, il Paese in cui l'indebitamento netto è cresciuto di meno a paragone con altri Paesi europei, come ci ha ricordato adesso il Ministro dell'economia. Ma noi siamo il Paese del quale non si è avuta politica anticiclica nel corso della peggiore crisi dopo quella del '29. potremmo oggi subire gli effetti negativi di scelte di rientro dai deficit pubblici e dalle politiche monetarie lassiste, di cui ieri non abbiamo potuto giovarci per rendere meno grave e meno pesante socialmente la crisi. Quanto alla politica delle entrate, voi avete saputo proporci, all'inizio della più grave crisi dal 1929, la detassazione degli straordinari, la *Robin tax* ed ora il terzo scudo fiscale in sette anni. Vorrei proporvi di ragionare anche a questo proposito in termini un po' più sistemici. In primo luogo, la pressione fiscale sul lavoro è troppo alta.

della capacità del Governo di trovare le risorse per la cassa integrazione in deroga nel corso di quest'ultimo anno di crisi! Sono anni, anni e anni che le imprese e i lavoratori italiani pagano molto di più in termini di contributi di quanto non ricevano per prestazioni da cassa integrazione. È possibile che non sappiamo nemmeno utilizzare questa occasione? Non ce l'abbiamo fatta noi come governi di centrosinistra, ma voi state facendo se è possibile persino peggio non utilizzando la crisi straordinaria che stiamo vivendo, almeno in questa chiave in una funzione positiva, per fare una riforma degli ammortizzatori sociali di tipo universale, giacché non è sostenibile dire che mancano le risorse necessarie. In ogni caso, tornando alla pressione fiscale sul lavoro, un riequilibrio graduale è possibile premendo di meno sul lavoro e di più sulle rendite. Se non si può o vuole farlo con l'unificazione al 20 per cento delle diverse aliquote oggi applicate ai redditi da capitale, allora si persegua lo stesso scopo portando le rendite nel reddito imponibile. I piccoli risparmiatori saranno tutelati e gli altri pagheranno come in altri Stati capitalistici. E tassiamo finalmente gli affitti con una aliquota unica del 20 per cento, accompagnata da una forte detrazione per l'inquilino. Secondo: a questo proposito, nella crisi abbiamo imparato che, grazie alle garanzie implicite fornite dagli Stati a spese dei contribuenti le grandi banche non possono fallire; è una buona notizia. E bene ha fatto il Governo italiano nei mesi scorsi, all'inizio della crisi, a mettere a disposizione le norme, le regole e le risorse necessarie per realizzare anche in Italia questa garanzia. Peccato che adesso il Ministro dell'economia stia autoriducendo l'effetto positivo di questa norma con una polemica sul mancato uso dei cosiddetti Tremonti *bond*, che a mio giudizio non sta né in cielo né in terra. Ma penso che, alla luce di quel che è accaduto, sia opportuno chiederci se non sia giusto che le banche paghino un piccolo premio per questa assicurazione, che nel corso della crisi è diventata un'assicurazione esplicita, ma che resta come assicurazione implicita anche quando quella esplicita venga ritirata. un piccolo premio, proporzionale alle dimensioni della leva finanziaria, pagato dalle banche a favore dello Stato, cioè dei contribuenti a carico dei quali si mette la garanzia di ultima istanza

che accresce i rischi sistemici, e spingerebbe le banche ad orientarsi al loro vecchio e buon mestiere: raccogliere soldi e prestarli alle imprese, riducendo le dimensioni di una leva finanziaria ingigantita dalla produzione di titoli che oggi tutti, "a babbo morto",

Si potrebbe dire che aumentano le spese e diminuiscono le entrate. Aggiungo che le entrate tributarie passano da circa 457 miliardi

come è stato ricordato anche oggi dal ministro dell'economia Tremonti, a che punto arriva. Tutti gli indicatori dicono che la crisi non è superata. C'è anche un altro indicatore, signor vice ministro Vegas, e riguarda le pensioni anticipate, che oggi fanno paura. Tra gennaio e luglio, gli assegni di anzianità liquidati sono stati 19.670 in meno rispetto alle previsioni ed a fine anno caleranno del 60 per cento rispetto al 2008. Cioè, la gente non va in pensione perché ha paura di questa crisi, che non è superata. Non è con l'ottimismo che si riescono ad affrontare e risolvere i gravi problemi del Paese!

seppellita sotto un buco di 3 miliardi di euro. Si tratta di banche, senatore Morando, che ai piccoli imprenditori

per cento previsto in primavera. Leggiamo tanti dati e neanche riusciamo a raccapezzarci.

che dicono cose molto diverse: il superindice OCSE riassume variabili mensili relative alle aspettative sulla fiducia delle famiglie e delle imprese. Come possiamo constatare, anche l'ISAE, che risponde al Ministero dell'economia, sostiene che la fiducia delle imprese è scesa; è migliorata leggermente quella delle famiglie, mentre quella delle imprese è scesa. Per l'Italia, il superindice dell'OCSE contiene sei voci: tre relative alle aspettative future (tra cui la fiducia delle famiglie e le aspettative delle imprese manifatturiere), dall'ISTAT e una dalla Banca d'Italia sul tasso d'interesse sul mercato interbancario a tre mesi. Molte di tali variabili sono incluse nel calcolo dell'indice degli altri Paesi OCSE. L'indice della Francia e del Regno Unito comprende anche il numero delle registrazioni di nuove automobili; quello francese considera anche il numero dei posti di lavoro vacanti. Rispecchiando l'elevata proiezione estera dell'economia tedesca e l'importanza del turismo per l'economia spagnola - stendiamo un velo pietoso sul turismo in in Italia - l'indice della Germania include il portafoglio ordini sull'estero. Il dato del PIL, quando esce, sembra una fotografia un po' datata del passato recente. Il superindice è invece una previsione basata sulle aspettative di chi opera nell'economia, si informa e segnala quando la situazione potrebbe iniziare ad andare meglio. I due indicatori mostrano andamenti differenti, il che è del tutto normale quando ci si avvicina alla fine di una recessione. Per ora è vero che l'Italia si avvicina a motore spento alla fine del tunnel, così come è anche vero che gli italiani sono ottimisti sul futuro, il che potrà contribuire a un più ravvicinato ritorno alla crescita nel nostro Paese. Resta comunque il fatto che né il superindice OCSE né altri indicatori possono dirci, con un ragionevole grado di affidabilità, quanto efficace sarà davvero la ripresa nel creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese. Posti di lavoro che sono falcidiati ogni giorno, perché ogni giorno chiudono fabbriche grandi e piccole. La cosa più probabile, semmai, è che il mercato del lavoro subisca ancora a lungo le conseguenze della crisi dell'ultimo anno. Per questo motivo non bisogna abbassare la guardia.

varato dal Governo italiano: «Utile nel breve periodo, rischia di rivelarsi dannoso nel lungo termine. Lo scudo», afferma Brian Coulton, responsabile per i *rating* europei di Fitch, a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale a Istanbul, «aiuterà il deficit, ma siamo un po' delusi dalla scelta di usare di nuovo

Coulton, «la ripetizione dei condoni mina la fiducia dei contribuenti» (quelli onesti, aggiungiamo noi) «e non incoraggia la cultura del pagamento delle tasse». Per questo egli è «preoccupato per gli effetti di medio termine» e sottolinea che lo scudo fiscale «non è una risposta fiscale ottimale per un Paese che ha problemi soprattutto sul versante della spesa». Al contrario, «può avere effetti dannosi nel lungo periodo, sebbene possa rivelarsi utile portare euro nel breve. Anche il ministro Tremonti», conclude Coulton, «ha perso un po' di credibilità su questo, perché aveva detto che non si sarebbe ripetuto». Ora, tutti sanno che l'Italia dei Valori ha condotto una battaglia contro questo condono, una battaglia molto forte perché è davvero

ha subìto la chiusura a tempo determinato per circa 20 giorni. Voi, invece, fate lo scudo per salvare i soliti furbetti del quartierino

manovra di aggiustamento delude anche le aspettative di quel terzo settore, di quelle associazioni di volontariato per le quali i contribuenti hanno versato il 5 per mille e che aspettano il pagamento per il 2007 e per il 2008. Invece del pagamento, poiché il Ministro dell'economia e l'Agenzia delle entrate credono che gli evasori fiscali siano nelle associazioni di volontariato, essi inviano questionari per rendere più difficoltosa la vita di queste associazioni. Non è questa la strada. Ce ne dispiace e siamo pertanto molto severi nei confronti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, secondo la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria che il Governo sottopone all'attenzione di quest'Aula, oggi saremmo in presenza di un miglioramento degli indicatori economici tale da far prefigurare per l'economia italiana uno scenario più favorevole rispetto al DPEF 2010-2013 per il biennio 2009-2010. Sembrerebbero insomma essere confermate le dichiarazioni di molti esponenti del Governo (in particolare del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e secondo i quali la crisi economica sarebbe già alle spalle e ciò renderebbe dunque non necessario né urgente operare pesanti interventi sull'economia italiana. In realtà, queste dichiarazioni sono semplici giustificazioni all'immobilismo del Governo, il quale tuttora non sembra in grado di approntare misure adeguate ad arginare le conseguenze della crisi. La situazione del mondo del lavoro costituisce la tragica prova di ciò. I dati statistici sull'occupazione, sia a livello internazionale che a livello nazionale, confutano infatti le visioni ottimistiche del Governo. L'analisi di tali dati, nella loro cruda semplicità, basta per capire come la situazione sia assai meno rosea di quanto si voglia far credere. Il Fondo monetario internazionale è stato chiaro: se la ripresa è iniziata, la crisi non è certo finita. Ci si troverebbe invece in quella fase economica assai pericolosa che viene definita *jobless* *recovery*. Saremmo cioè in una situazione di ripresa senza lavoro. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'istituto di Washington, il tasso di disoccupazione in Europa nel 2009 si attesterà al 9,6 per cento e nel 2010 sarà addirittura dell'11,7 Per quanto concerne specificamente l'andamento dell'occupazione in Italia, basterebbe riportare testualmente quanto scritto dall'ISTAT nella rilevazione sulle forze di lavoro del secondo trimestre 2009: «L'offerta di lavoro registra, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione di 241.000 unità. (...) Nel secondo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (-1,6 per cento, pari a -378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei dipendenti a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori». Non certo di segno diverso sono i dati pubblicati sempre dall'ISTAT su lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese e i dati diffusi dall'INPS relativamente al ricorso alla cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria. Le cifre lasciano poco spazio ai dubbi: fra il settembre del 2008 e l'agosto del 2009, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'INPS ha registrato un aumento del 53 per cento delle domande di indennità di disoccupazione. Il totale delle richieste avrebbe raggiunto quota 1.100.000, di cui sarebbero oltre 984.000 quelle ammesse. Se è vero che, come precisato dallo stesso istituto di previdenza, il rapporto tra richieste e beneficiari è di circa uno a due (cioè due richieste per ciascun lavoratore) è comunque possibile stimare che alla fine dell'anno 2009 i disoccupati in Italia saranno circa 500.000. In tal senso vanno anche le previsioni formulate dal Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro. I numeri della cassa integrazione guadagni sono parimenti spaventosi. Per quanto concerne la cassa integrazione ordinaria, essa è aumentata del 409 per cento, mentre la straordinaria sarebbe aumentata dell'86,7 In questa situazione già di per sé drammatica sono ben 200.000 i lavoratori che vedono avvicinarsi la scadenza delle 52 settimane previste dalla legge per la cassa integrazione ordinaria. Nel complesso, il Fondo monetario internazionale prevede per l'Italia a fine 2009 un livello di disoccupazione pari al 9,1 per cento, con un aumento fino al 10,5 per cento Il fatto che tale dato sarebbe al di sotto della media europea non serve certo di conforto alle migliaia di lavoratori a rischio o che hanno già perso il posto di lavoro. Il Governo conosce perfettamente i dati contabili e statistici. E come affronta la situazione? Con l'oscuramento mediatico dei problemi del lavoro o con una guerra alle organizzazioni sindacali più attente. Dall'esame di questo Documento e della legge finanziaria 2010 non giungono risposte. Di fronte a quasi 400.000 posti di lavoro persi nel secondo trimestre del 2009, il Governo non sembra avere nessuna cura efficace da proporre. Presenta una finanziaria che è stata definita leggera, un provvedimento che da un lato è la spia evidente della mancanza di idee su come affrontare le conseguenze della crisi economica e dall'altro sembra essere l'ennesimo provvedimento-manifesto volto a tranquillizzare gli animi. Tra l'altro, presenta anche aspetti grotteschi, come l'indicazione dell'Atto Senato n. 1167, il cosiddetto collegato lavoro alla finanziaria 2009 e non ancora approvato, come collegato alla finanziaria 2010. Altre e più urgenti sembrano essere le priorità di questo Governo. E nessuna di esse riguarda il lavoro. Eppure, paradossalmente, questa crisi offre un'occasione per intervenire sulla squilibrata situazione italiana, cui vi sono categorie di lavoratori che godono di alcune forme di protezione (nell'industria, nella distribuzione commerciale con oltre 50 dipendenti e nelle imprese di servizi con più di 200 dipendenti) e altre (i dipendenti delle imprese più piccole,

il Governo sta centellinando le erogazioni comportandosi come se non ci fossero soldi sufficienti. In realtà, solo la cassa integrazione guadagni ha un bilancio attivo stimabile in 10 miliardi di euro. È il momento di utilizzare questa grande quantità per porre mano ad una vera riforma degli ammortizzatori sociali, creando un sistema universale di indennità di disoccupazione che assicuri a tutti i lavoratori rimasti senza lavoro il trattamento pari all'80 per cento della retribuzione. È il momento di porre in essere una seria e generale politica di lotta alla disoccupazione, con particolare attenzione al Mezzogiorno. È il momento di operare per la riduzione della pressione fiscale, a partire dal mondo del lavoro, attraverso un aumento della detrazione IRPEF per lavoro dipendente, una riduzione del prelievo fiscale sulla quota di salario dovuta agli aumenti del rinnovo dei contratti di lavoro, una detassazione delle tredicesime È il momento di agire, di dare risposte adeguate ai cittadini italiani, e non di attendere di fare cassa con il rientro dei capitali

finestra") *(PdL)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, vice ministro Vegas, onorevoli senatrici e senatori, siamo giunti al capolinea delle Note di aggiornamento, se anche l'altro ramo del Parlamento approverà la riforma della finanza pubblica per cui dal prossimo anno il

ma del complesso delle previsioni per la definizione del bilancio dello Stato. Non è inopportuno - anzi è dovere del Parlamento - in momenti come

Infatti, si deve osservare che le condizioni eccezionali dell'economia e della finanza pubblica e privata, come conseguenza degli effetti della crisi mondiale, rendono l'esigenza di questo aggiornamento delle previsioni propedeutico al varo della legge finanziaria e del bilancio di previsione annuale e triennale che affronteremo durante questa le variazioni intervenute nell'arco dell'ultimo trimestre nel quadro previsionale sono infatti tali da modificare in modo sostanziale le prospettive della finanza pubblica. In particolare, il miglioramento della congiuntura internazionale ha visto un immediato riflesso sull'andamento dell'economia italiana nel corso dei mesi estivi; anzi, il nostro Paese, secondo l'indicatore anticipatore della congiuntura elaborato dall'OCSE, ha una delle migliori *performance*, seguito dalla Francia tra gli altri Paesi più industrializzati. I dati macroeconomici trovano riscontro nelle statistiche che determinano il grado di fiducia dei consumatori. In parte sono state citate nell'intervento di oggi del Ministro dell'economia: si dà un indice del 113 rispetto al precedente 111 di agosto; quindi, segni di recupero vengono da varie indicazioni da parte dei centri di studio: studio: per la prima volta, dal marzo 2002, un indicatore complessivo con un saldo positivo. Questo, lo vorrei dire, perché c'è un dato a mio avviso fondamentale: abbiamo sentito nelle varie relazioni gli spostamenti - lo 0,2, lo 0,3 - rispetto alla previsione precedente e le altrettante previsioni che valutano su decimali di punto. Io ritengo però che l'indicatore dello stato d'animo, se positivo, in un'economia di mercato come quella dei Paesi occidentali, che ha il motore del suo vivere non sul puro stato di bisogno primario ma su una condizione di attesa e di aspettativa,

Anche basandosi su tale previsione di miglioramento e sui risultati già conseguiti nel secondo trimestre del 2009, la Nota di aggiornamento ritiene che la diminuzione del PIL sarà più contenuta rispetto a quanto indicato nel mese di luglio: passiamo dal 5,2 al 4,8, e anche in questo caso occorre osservare che le previsioni dei diversi istituti si rincorrono in queste settimane e tutte sembrano segnare un costante aggiustamento delle indicazioni in miglioramento rispetto a quelle precedenti. Analogamente, si prevede nel 2010 una leggera ripresa, con una previsione di crescita dello 0,7 per È apprezzabile come il Governo, prudenzialmente, abbia tenuto comunque sul triennio 2011-2013 una crescita del PIL che si attesta sul due Le note di maggiore criticità della Relazione previsionale e programmatica riguardano l'andamento occupazionale. Già altri colleghi hanno voluto citarlo: il mercato del lavoro sconta un ritardo di circa un semestre rispetto all'andamento economico congiunturale, per cui, al di là dell'incertezza sull'effettivo impatto, si può ritenere che, allo stato attuale, la situazione dell'occupazione possa essere ancora soggetta a ulteriori ridimensionamenti. C'è comunque da rilevare che l'Italia è, tra i Paesi europei, quello che ha avuto effetti più contenuti sul mercato del lavoro, e ciò anche grazie all'intervento massiccio con gli ammortizzatori sociali. Appare però comunque inevitabile che una quota di occupati, che oggi beneficia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, sia sostanzialmente destinata a incorrere nel meccanismo degli esuberi, in considerazione del fatto che che anche la ripresa porrà alle imprese il problema di ristrutturare la propria organizzazione in funzione delle nuove opportunità, naturalmente puntando sul recupero della produttività per essere più competitivi; purtroppo, però, la ripartenza dei treni non aggancerà tutti i vagoni.

compensata però dall'atteso peggioramento del saldo primario. Per il 2009 c'è la conferma dell'incidenza dell'indebitamento netto sul PIL al 5,3 per cento, scontando quindi un miglioramento in valore assoluto sul saldo di bilancio.

Questo è uno dei momenti in cui è necessario valutare gli effetti permanenti dei provvedimenti anticrisi sui conti pubblici e, naturalmente, anche l'effetto del raggiungimento del 115 per

ma si può pensare di fermarne la crescita e naturalmente, a questo punto, cominciare a cambiare

vorrei tentare di fare una sintesi rispetto delle tante cose importanti che sono state dette nel corso di questa discussione. Nella Nota di aggiornamento 2010-2013, almeno dal nostro punto di vista, l'unico dato certo che abbiamo è che, se il Governo ha l'obbligo di presentare il DPEF e la Nota di aggiornamento per consentire alle Camere di esaminare i contenuti e definire l'entità della successiva manovra finanziaria e le ripercussioni che essa avrà sui saldi di finanza pubblica (e quindi, per capirci, non parliamo di indicazioni di carattere semplicemente programmatico, ma di decisioni che assumono un rilievo vincolante per la successiva sessione di bilancio), allora anche questa Nota, come il precedente DPEF, disattende palesemente la legge di contabilità. Resta l'assenza, direi colposa, di una articolazione degli interventi necessari per gli obiettivi prefissati e, soprattutto, come prescrive la legge 5 agosto 1978, n. 468 (che è ancora in vigore), resta l'assenza di una valutazione di massima dell'effetto economico‑finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale. Di fatto, si conferma che la direzione intrapresa dal Governo continua a essere più il frutto di aggiustamenti progressivi e di tentativi spesso annunciati e poi messi da parte, piuttosto che un percorso chiaro dai confini ben delineati. Per il periodo che viviamo, signor Vice Ministro, ci saremmo attesi ben altro, proprio sul merito e sull'entità delle scelte, perché queste ultime nei prossimi mesi saranno - e lo vedremo il vero terreno di confronto, né facile né scontato, sia con le parti sociali, sia con gli enti locali, ma stiamo vedendo anche, e soprattutto, all'interno dello stesso Governo. Quel che è certo è che si continua a non fare nulla per accelerare l'uscita dalla crisi e per renderla più accettabile sul piano sociale e più sopportabile sul piano umano: tre posti di lavoro su quattro sono distrutti dalla crisi, e si tratta di contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate, lavori atipici, tutte posizioni non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali (quelli, per intenderci, considerati dal Ministro del lavoro i migliori del mondo). Non ci sono risorse aggiuntive per gli ammortizzatori in grado di coprire quel mezzo milione di persone che ha già perso il lavoro e che è stato fin qui ignorato. Non ci sono le riduzioni delle tasse sul lavoro e neanche i grandi piani per lo sviluppo del Mezzogiorno annunciati subito dopo aver finto di cedere 4 miliardi alla Regione Sicilia. Non ci sono fondi per la ricerca e l'università e non c'è una spinta alla nostra economia che sarebbe dovuta arrivare, come era stato detto, anche dalle nuove regole della contrattazione.

ci troviamo di fronte a numeri e non a conti e resoconti delle misure messe in campo per fronteggiare la crisi. Quindi, più che a una fotografia del bilancio dello Stato, come è stata definita dal ministro Tremonti, ci troviamo di fronte a un disegno confuso e sbiadito, fatto di dati discordanti ai quali volutamente non si vuole dare una lettura realistica. E qui, sia chiaro, non si tratta, come ha sentenziato in modo un po' sprezzante il Capo del Governo, dell'opposizione che è anti-italiana perché fa il tifo per la crisi economica: si tratta di non accettare l'incompletezza e la cosciente genericità dei dati contenuti in questa Nota e nel DPEF di luglio. Partiamo dai dati del PIL, la cui decelerazione di caduta è stata presentata come un segnale positivo. In realtà, ci si è guardati bene dal rilevare che il dato cumulativo, dal secondo trimestre del 2008 al secondo trimestre del 2009, è peggiore di tutti gli altri Paesi del G20, e solo il Giappone ha sin qui fatto peggio dell'Italia. Non è certo migliore il quadro previsionale relativo al mercato del lavoro perché, se da un lato si evidenzia il miglioramento degli indicatori economici del superindice OCSE, dall'altro si sottace l'analisi dell'impatto della recessione, anch'essa - guarda caso - recentemente pubblicata nell'Outlook dell'OCSE, dove, sulla base dei dati disponibili, si evidenzia che alla metà del 2009 la maggior parte dell'incremento atteso dell'occupazione ha preso piede in Irlanda, Spagna e Stati Uniti, mentre in altri Paesi, come l'Italia, la gran parte di tale incremento deve ancora avvenire.

il dato preoccupante è che al Sud non c'è corrispondenza tra persone licenziate e chi è in cerca di nuova occupazione. È un segnale sconfortante, in quanto aumenta la popolazione inattiva di chi non cerca un lavoro perché sa di non poterlo trovare e di chi a volte si rifugia nell'unica possibilità offerta dal mercato, che è il lavoro nero. Sul lato della spesa nell'anno 2009 si conferma una accelerazione della spesa corrente al netto degli interessi, al cui interno continuano a nascondersi sprechi, inefficienze, problemi non risolti, spesa che giunge ai livelli record del 43,1 per cento, mentre negli anni successivi si riduce drasticamente in termini nominali la spesa in conto capitale e la spesa per gli investimenti. Ma anche qui le cifre sono del tutto parziali e in parte - consentitemi, con rispetto parlando - taroccate. Per valutare la tenuta delle previsioni, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse fornito elementi relativi agli esiti dei tavoli di verifica e monitoraggio e soprattutto alle prospettive per la sanità sanità alla luce della prossima intesa Stato-Regioni. Né il Ministro dell'economia, né quello della salute hanno dato sinora risposte convincenti agli interrogativi che sono stati sollevati dalle Regioni e che hanno posto un problema semplice, ma anche molto serio: prima di tutto bisogna discutere sulle risorse destinate al Fondo nazionale per la sanità e a quello per la non autosufficienza, perché si tratta di una dote, quella proposta, insufficiente a garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza. E se il Governo vuole ridurre ulteriormente gli stanziamenti, se ne dovrà assumere sino in fondo e per intero ogni responsabilità. Appare poi poco credibile la riduzione di spesa per prestazioni sociali negli anni successivi al 2009, come prevista nella Nota di aggiornamento, se queste spese sono riconducibili non solo all'aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore pubblico, ma soprattutto all'attesa di migliori prospettive di occupazione che così comporterebbero un minore ricorso alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali. Si capisce come le attese potrebbero essere facilmente disattese. Sarebbe stato infine utile e necessario che il Governo avesse fornito un quadro dettagliato sull'articolazione delle misure *una tantum*, dei loro effetti, della loro efficacia con l'analisi dei saldi strutturali. Se analizziamo le misure anticrisi per tipologia di intervento vengono fuori delle sorprese sottaciute o omesse. Nel sostegno al settore industriale, alle imprese, le risorse messe in campo (quasi la metà di quelle complessive) dovevano finanziare principalmente interventi volti a facilitare l'accesso al credito e ad allentare i vincoli di liquidità per le piccole e medie imprese, mentre in realtà il credito alle imprese si sta contraendo. Il differenziale nel costo del credito tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord si è nuovamente ampliato nel primo trimestre di quest'anno e le banche non sembrano affatto essere attratte dal sostegno pubblico con i Tremonti *bond*, che considerano un buon affare solo per il Tesoro. Nelle misure volte a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro - e tra queste rientra il finanziamento degli ammortizzatori sociali - sono preoccupanti, alla luce dei dati di di cui parlavamo poc'anzi, le affermazioni del ministro Sacconi, secondo cui per gli ammortizzatori sono stati spesi solo 1,5 miliardi di euro sugli 8 preventivati e stanziati. Se non ora, quando?

sostanzialmente in un *bonus* straordinario, *una tantum*, per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, che per l'esiguità dell'importo ha prodotto e produrrà effetti assai modesti. Per queste ragioni, prendendo atto dell'inesistenza di qualsiasi seria reazione alla crisi in atto, dell'inesistenza di una politica economica nazionale, di una strategia nazionale di contrasto al deterioramento dell'economia, vogliamo impegnare il Governo, con la nostra risoluzione, a riformulare la Nota di aggiornamento 2010-2013, perché si devono e si possono introdurre specifiche indicazioni aggiuntive. Noi le riassumiamo in una estensione e rafforzamento degli ammortizzatori sociali, in una riduzione e redistribuzione della pressione fiscale, in un maggiore controllo sulla dinamica delle imposte indirette e, infine, in una visione unitaria del Paese che sia a salvaguardia di un'azione di riduzione del divario tra Nord e Sud. Di tutto questo, secondo noi, ha bisogno il Paese e riteniamo che non sia più consentito sul piano economico, politico ed etico l'alibi di ulteriori ritardi Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione